Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"

Signor Presidente, il presente disegno di legge è volto alla ratifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. L'accordo che si sottopone all'*iter* parlamentare di ratifica oggi, tenuto conto dell'attuale contesto economico e di mobilità tra l'Italia e la Svizzera, definisce il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri. In merito agli aspetti generali, si evidenzia che le disposizioni dell'accordo prevedono innanzitutto il principio di reciprocità. A differenza del precedente accordo del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, il presente accordo disciplina anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia. Quanto al metodo di imposizione, l'accordo stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'80 per cento di quanto dovuto dallo stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato. L'accordo fornisce una definizione di aree di frontiera, nonché una definizione di lavoratori frontalieri e prevede inoltre alcune disposizioni transitorie relative agli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera, ai quali si applica il regime di tassazione esclusiva in Svizzera. L'accordo comprende dieci articoli e un Protocollo aggiuntivo. PRESIDENTE.

Signor Presidente, ha già detto tutto il collega Borghesi. Voglio solo integrare dicendo che, mentre nel 1974 l'Accordo tra Italia e Svizzera era unilaterale e quindi si riferiva esclusivamente ai lavoratori italiani che andavano in Svizzera, quello che trattiamo oggi, come ha detto correttamente il senatore Borghesi, ha invece un carattere di reciprocità, il che significa che vale anche per i lavoratori svizzeri che vengono in Italia. Credo sia giusto rimarcare questo aspetto, perché è un indice chiarissimo del fatto che la situazione economica nei territori limitrofi al confine svizzero si sia evoluta in maniera positiva per il nostro Paese. Per il resto mi rimetto a quanto detto dal collega Borghesi.

vengono poste le basi per la sottoscrizione di questo nuovo accordo fiscale: ai tempi c'era il Governo Renzi, così almeno ci chiariamo bene.

vengono coinvolte anche la Province di Varese, di Como e di Sondrio, i sindacati, le Camere di commercio e tutte le associazioni proprio per cercare di elaborare delle proposte che tendano a migliorare l'accordo. E dove si arriva?

prevede che le risorse maggiori incamerate dallo Stato a seguito della nuova imposizione possano essere usate per dare sostegno ai Comuni che si trovano nell'area di confine.

abbia la Regione e sostenendo che questa sia una competenza prevalentemente statale. Occorre però tenere presente che, in fase di proposta, le Regioni interessate possono assolutamente lavorare e creare delle condizioni, proprio per avanzare proposte che vanno in questa direzione.

Quindi era giusto sottolinearlo, perché di questa volontà di appropriarsi sempre dei meriti altrui siamo abbastanza stanchi e quindi vorremmo essere un po' più precisi e dire le cose come stanno. C'è però di più - e mi avvio a concludere

legge, per realizzare infrastrutture e servizi per le zone di confine, possa essere utilizzato anche

un principio che va proprio nella direzione delle zone economiche speciali, perché aumentare i salari per quelli che lavorano nelle aree di confine è naturalmente un primo segnale importante che finalmente il Governo e lo Stato italiano nei confronti di queste zone che vivono una situazione di fortissima difficoltà e che spesso sono state tenute in scarsa considerazione da tanti Governi che si sono succeduti negli ultimi

che non a caso, dal punto di vista della tecnica legislativa, esula rispetto alla modalità tradizionale con la quale il Parlamento è chiamato a dover ratificare dei trattati internazionali. In genere, anzi sempre, nei percorsi di ratifica internazionale noi siamo chiamati ad approvare il testo dell'accordo sottoscritto fra i singoli Governi senza entrare nel merito, nel merito, perché così prevede la normativa, e sostanzialmente molto spesso senza entrare all'interno di una discussione politica rispetto a questi contenuti. In questo caso, invece, siamo in presenza sia di una discussione nel merito degli accordi, sia di una serie di norme di accompagnamento che vigono sul regime impositivo interno, in questo caso italiano, che costituiscono un importante avanzamento del sistema dei diritti e delle garanzie per molti lavoratori italiani, che ogni giorno si recano nella Confederazione elvetica per lavorare. Come correttamente e opportunamente ha ricordato all'Aula il relatore Spagnolli, ciò avviene anche in un principio di reciprocità, per cui per la prima volta anche i lavoratori svizzeri che vengono in Italia vengono sottoposti ad uno specifico regime giuridico. inserisca all'interno di un contesto particolare ce lo dicono i dati. Presidente, molto spesso il tema del rapporto con la Svizzera viene derubricato a marginale o periferico; in realtà i numeri ci dicono l'importanza di una relazione di questa natura, non solo perché la Svizzera è il Paese con il quale abbiamo la frontiera più estesa (740 chilometri), non solo perché gli investimenti svizzeri in Italia ammontano a 16 miliardi, non solo perché la Svizzera è il sesto Paese di destinazione per l'*export* italiano e conta come la Cina e l'India insieme, non solo perché in quindici anni l'Italia ha totalizzato più di 39 miliardi di euro di surplus

ogni giorno più di 70.000 italiani, 68.000 dei quali residenti in alcune Regioni confinanti, si recano a lavorare all'interno di questo territorio straniero straniero e abbisognavano di una ammodernamento dello strumento giuridico. Questo anche in considerazione di una serie di prese di posizione che vi sono state negli anni scorsi, quando, a fronte di una proposta di sovranismo ticinese, svizzero, che vedeva sui lavoratori italiani addirittura scaricare una campagna di stampa culturale e politica

condotto dall'allora vice ministro e oggi nostro collega di Gruppo, senatore Antonio Misiani, che seppe svolgere un'attenta azione di ascolto e di concertazione con i territori, con le parti sociali e con tutti gli *stakeholder* interessati, per raggiungere alcuni obiettivi significativi, che provo molto rapidamente a enucleare. anzitutto sancito un principio fondamentale in una nostra legge, che assicura anche un po' di pace all'Agenzia delle entrate, che ogni volta interpreta in maniera un po' singolare questi lavoratori: all'articolo 3 si sancisce che i lavoratori frontalieri residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera. Questo potrebbe sembrare pleonastico, ma fino a questo momento non c'era alcuna norma che lo sancisse e questo dava adito molto spesso a una serie di interpretazioni un po' singolari dell'Agenzia delle entrate. Viene estesa la franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri, che viene a portata 10.000 Viene introdotto il meccanismo relativo ai redditi prodotti dai lavoratori frontalieri svizzeri in Italia e, soprattutto, vengono introdotte una serie di norme sia a garanzia dell'attuale gettito che i lavoratori frontalieri garantiscono ai Comuni di frontiera, sia in termini di assicurazione rispetto al fatto che il futuro gettito che deriverà dall'applicazione di questo accordo

prevede un particolare meccanismo, il cosiddetto meccanismo dei ristorni, che consente una serie di gettiti a favore dei Comuni di frontiera. L'introduzione originaria di una diversa modalità avrebbe potuto comportare l'eliminazione di questi fondi. Invece grazie al nostro lavoro, in particolare grazie al lavoro del Partito Democratico e del Governo del quale abbiamo fatto parte, questo gettito viene garantito ed è cifrato in termini di 89 milioni, che è il valore più alto rispetto al precedente anno di applicazione (2019) di questo tipo di accordo. gettito verrà portato fino in fondo attraverso un meccanismo di garanzia statale. Quindi i Comuni di frontiera non hanno nulla a che temere dall'introduzione di questa Il secondo aspetto particolarmente significativo è il fatto che il gettito in aumento progressivo derivante dall'applicazione del nuovo regime dei lavoratori frontalieri, che avverrà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla ratifica, anche in questo caso assicurando che gli attuali lavoratori non vedranno in alcun modo modificato il loro regime fiscale e il loro regime previdenziale, andando incontro a una serie di esigenze e di prospettive che ci sono state rappresentate sui territori, dicevo il maggiore gettito derivante dall'applicazione del nuovo regime fiscale ai nuovi lavoratori frontalieri verrà mantenuto sui territori originari. È questa una prima prova

di progressiva applicazione di questa normativa, di creare un fondo per le infrastrutture e lo sviluppo economico delle zone di confine italo-elvetiche, che parte con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2025, per arrivare a regime a 221 milioni nell'anno 2045. Presidente, che chiederemo di intervenire sull'emendamento annunciato dal collega Romeo, in quanto vi sono una serie di elementi e di tecnicismi che richiedono, dal nostro punto di vista, una puntualizzazione. In ogni caso, questo elemento consente di assicurare, così come previsto da un ordine del giorno approvato nel 2017 su proposta del Partito Democratico, che le zone di confine abbiano un loro specifico fondo di sviluppo. Ciò a dimostrazione del fatto che, quando si lavora in

l'importante elemento finale di questo disegno di legge è l'istituzione di uno specifico tavolo interministeriale, al quale tutti i soggetti dedicati a questo tipo di a questo tipo di prerogativa saranno chiamati al fine di discutere delle proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro, dialogo sociale e cooperazione transnazionale per la definizione di uno statuto dei lavoratori frontalieri. È un tema che fino adesso non aveva mai avuto nessuna copertura giuridica, che aveva fatto sì che questi lavoratori rimanessero in un limbo giuridico, politico e culturale; un limbo dal quale questa legge li trae, per dare loro quella giusta dignità, quella giusta garanzia che spetta a loro in un quadro di tenuta delle relazioni istituzionali tra Italia e Svizzera, in una prospettiva di integrazione e di lavoro comune.

il ricorso al telelavoro da parte dei lavoratori frontalieri con modalità più ampie e più agevoli. Vi era un accordo amichevole, che però, dal 1° febbraio 2023, cioè da

quando il Vice Ministro dell'economia e delle finanze era il collega Misiani, a prendere atto di una situazione che si era creata nei territori di confine, dove molte aziende ricorrevano allo *smart working* proprio per far fronte all'emergenza Covid-19. Costruimmo un accordo amichevole, che permetteva, anche a coloro che trascorrevano più del 25 per cento delle giornate lavorative rimanendo in Italia, nelle fasce di confine e non solo, di non essere tassati interamente in Italia con una penalizzazione molto forte sullo stipendio.

Le stesse imprese hanno capito tre cose: innanzitutto che potevano risparmiare sulle missioni, quindi non c'era bisogno di spendere tanti soldi perché l'alfabetizzazione digitale che abbiamo fatto in quel periodo ha portato a utilizzare molto di più le *video call*, tutti i sistemi e le piattaforme che permettevano di farlo; in secondo luogo, che risparmiano sugli affitti perché affittano immobili meno grandi e quindi utilizzano in maniera più estensiva

ieri questo accordo amichevole. Pensiamo che invece si debba continuare a farlo sulla base di nuove motivazioni,

alla Camera che vanno in questa direzione; il Governo ha mostrato un'apertura, però bisogna fare in fretta perché l'Agenzia delle entrate nel frattempo ha già mandato messaggi molto chiari ai contribuenti lavoratori frontalieri che devono pagare le tasse in Italia con una notevole penalizzazione. Quindi, è bene che il Governo faccia in fretta.

L'ordine del giorno era quello che avevo annunciato in Commissione: la nostra intenzione era di presentare un ordine del giorno con il relatore o di tutta la Commissione affinché - come dice il senatore Romeo nessuno si appropriasse di meriti altrui e ci fosse un'unità di intenti per risolvere la questione. Come già accennato il senatore Alfieri, il Governo non è stato molto attento e ha fatto scadere questo accordo. Chi, come me e i cittadini lombardi, in queste settimane è stato in campagna elettorale nei luoghi quali Varese, si è accorto che la prima domanda che fanno i giornalisti è quella: ma lo *smart working*?

la dizione e ampliarla affinché venisse evidenziato che comunque si tratta di telelavoro, ma effettuato in un luogo diverso. Veniva meno così la necessità di cambiare le prassi e anche la tassazione, mitigare la risposta all'interpello di un cittadino dell'Agenzia delle entrate. Invitiamo il Governo a tenere conto di questa nuova definizione di lavoro da remoto e non di telelavoro come ampliamento e nuove possibilità di attuazione dell'accordo amichevole. i pareri sono favorevoli con le integrazioni e le modifiche decise a livello di Commissione e in accordo col Governo.

nei termini di seguito indicati: «Impegna il Governo ad adottare tutte le misure di propria competenza, al fine di avviare con urgenza negoziati con il Governo della Confederazione svizzera, volti a disciplinare il ricorso al telelavoro da parte dei lavoratori frontalieri, in ragione dell'imminente scadenza del precedente Accordo amichevole.».

esprimo parere favorevole a condizione che il dispositivo sia riformulato nei termini di seguito indicati: «Impegna il Governo a valutare l'opportunità, tenuto conto del numero di beneficiari dell'assegno unico, di adottare ogni iniziativa utile, al fine di accelerare la trasmissione da parte dell'INPS del modulo richiamato in premessa, nonché al fine di introdurre un meccanismo di autocertificazione degli importi.».

lavoro da remoto a telelavoro. Con questa riformulazione - secondo me - si va a restringere un po' il campo dell'operazione. Quindi, se fosse possibile, mantenere la definizione data attualmente - secondo noi - sarebbe più accettabile. Diversamente lo accogliamo comunque, ma

Signor Presidente, verrebbe da dire che siamo in presenza dell'ordinaria follia della burocrazia italiana. A seguito di una importante normativa che è stata introdotta nel nostro Paese nel corso della scorsa legislatura, e cioè l'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, abbiamo assistito a un'implosione interna all'INPS, che non ha trasmesso la documentazione relativa alle casse previdenziali svizzere. Il risultato è che i lavoratori frontalieri non possono più disporre del pagamento dei cosiddetti assegni familiari. E questo evidentemente -da una parte - conculca il loro diritto e - dall'altra - determina una serie di problematiche. È facilmente intuibile quali possano essere le conseguenze di un mancato pagamento e di un mancato introito determinato da misure di questa natura. Affinché la Svizzera possa erogare la differenza tra l'assegno elvetico e quello già erogato in Italia dall'INPS come ho detto - le casse di compensazione svizzere richiedono alle strutture INPS competenti per territorio di residenza la compilazione di un modulo specifico che si chiama E411. E la procedura di trasmissione di questo modulo

affinché sia possibile sbloccare questa situazione. La risposta del Governo è quella classica che "valuterà l'opportunità di". Vorrei darle una comunicazione, signora Sottosegretario: qui non c'è da valutare, qui c'è da lavorare,

accolga questo ordine del giorno nella sua formulazione originaria. Nel caso in cui si dovesse permanere nella occhiuta e burocratica dizione della valutazione, naturalmente - come si dice dalle nostre parti - piuttosto che niente è meglio piuttosto. Ma sicuramente continueremo a incalzare il Governo perché non sia una palla buttata in *corner*, perché i cittadini coinvolti attendono una risposta che il Governo deve dare.

Senatore Garavaglia, ho un'ulteriore richiesta da farle. Siccome, come avrà visto, c'è un parere condizionato della 5a Commissione, le chiedo se lo

Chiedo ai colleghi un momento di pazienza perché abbiamo una questione tecnica da sistemare.

Quello che può sembrare un costo in realtà non lo è. Si tratta, bensì, di un investimento: prevedere che, tra le finalità del fondo dei Comuni di confine, ci sia quello di integrare i salari per chi lavora alla frontiera nella parte italiana,

Allo stesso modo, dando dei premi a chi resta nel nostro territorio, si evita la chiusura di aziende e lo Stato continua ad avere lavoratori che versano le imposte. In questa ottica penso sia chiaro anche il senso di questo emendamento, che mi auguro venga accolto.

disattiva)* ..un'esigenza. Si ricordava prima il tema dello sconto benzina e della particolarità della specificità della fascia di confine dei venti chilometri. Noi dobbiamo restituire una parte di quelle risorse al territorio: esportando lavoratori e importando consumatori c'è un effetto di spiazzamento rispetto alle imprese che fanno fatica a individuare e a selezionare personale che faccia lo stesso tipo di lavoro che è pagato in modo migliore dall'altra parte del confine. Da questo punto di vista abbiamo l'esigenza sicuramente di dare una risposta sul versante al costo del lavoro, ma anche di costruire infrastrutture e mettere in campo progetti di sviluppo socioeconomico. I Comuni di quella fascia di confine non sono in grado, addirittura, a volte di prevedere l'addizionale Irpef, perché sarebbe estremamente discriminante che la popolazione che

di secondo livello sindacale, trovando dei meccanismi di coinvolgimento delle forze sociali per utilizzare una parte di tali risorse perché gli enti locali non possono dare risorse direttamente a quei lavoratori. Si tratta quindi di una questione delicata.

ci fosse la questione dell'«anche» e «non interamente sostitutivo». Chiedo solo conferma che sia effettivamente così. A me avevano assicurato una riformulazione di questo tipo: non più il discorso sostitutivo, ma ma la parte legata agli enti locali, che chiaramente vogliono intervenire e viene, quindi, salvaguardata la loro autonomia di intervento, avendo anche la possibilità di far sì che si possa utilizzare l'integrazione salariale. Questo è indubbiamente un principio, come detto prima. Chiedo quindi solo conferma che effettivamente si tratti di quanto mi è stato assicurato.

viene aggiunto al potenziamento delle infrastrutture il sostegno dei salari, rimandando alla questione che prima ha sottolineato il senatore Alfieri. È evidente che il sostegno dei salari è una competenza legata alla competenza statale e poi alla contrattazione di primo e secondo livello. È un elemento importante questo da dovere rimarcare. Non è una competenza degli enti locali, a cui originariamente veniva assegnato il fondo infrastrutturale. Quindi è un'estensione, ma anche un impegno successivo rispetto a una competenza di natura statale.

dichiarazione di voto. Fermo restando che come Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo votato a favore e voteremo a favore dell'Accordo in esame, vorrei che si evitasse di fare campagne elettorali in questo momento in Parlamento.

ad esempio, sul fatto che negli ultimi anni in Italia non basta lavorare per essere considerati fuori dalla povertà. Oggi anche un lavoratore rischia di essere povero. Ci sono lavoratori e lavoratrici che non riescono a progettare il futuro. Vorrei che la discussione sulle condizioni di lavoro questo Parlamento la facesse fino in fondo. È davvero facile discutere

di altri lavoratori, non dico frontalieri. Ora siamo di fronte a un fenomeno particolare, che conosco bene, avendolo seguito in parte quando ero sindacalista.

il decreto-legge aiuti *quater* e via dicendo, ma non abbiamo affrontato il fatto che i salari e gli stipendi dei lavoratori italiani stanno perdendo ogni giorno potere d'acquisto. È necessario individuare un meccanismo che sia in grado di adeguare

nelle due direzioni. Esprimo la soddisfazione del nostro territorio per aver raggiunto questa nuova regolamentazione, che sicuramente favorisce i lavoratori. Per il resto, mi rimetto a quello che ho detto in veste di relatore del provvedimento.

parte della paternità della negoziazione sugli accordi. Ma la verità è che quello di oggi è un atto dovuto per 90.000 lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, che, in assenza di accordo, si troverebbero a vedere applicato quello che l'Agenzia delle entrate ha deciso con un interpello. Quindi, forse, per una volta possiamo essere orgogliosi del fatto che una tale risposta è un atto dovuto per quei lavoratori. Il disegno di legge di ratifica, che oggi esaminiamo nel testo unificato dei disegni di legge 108, a prima firma Alfieri, e 376 del Governo, approvato dalle Commissioni riunite 3a e 6a, riguarda la ratifica degli accordi tra Italia e Svizzera siglati nel dicembre 2020 e già ratificati con il voto parlamentare dello scorso 26 gennaio.

di riflessione. È vero che c'è il tema del telelavoro, che bisogna disciplinare; è vero che c'è il tema dello *smart working* e delle modalità in cui si organizzano le prestazioni lavorative, oggi in maniera diversa a prescindere da quello che è stata l'emergenza dovuta alla pandemia,

a tutte le altre situazioni di lavoratori frontalieri riguardanti altri Paesi confinanti. Prima il senatore Spagnolli ricordava che oggi noi stiamo parlando dei frontalieri italo-svizzeri, ma abbiamo temi simili che riguardano altri territori. Ricordo, per esempio, un ordine del giorno a prima firma della senatrice Paita che chiede di promuovere un percorso di aggiornamento degli accordi relativi ai lavoratori frontalieri di altri Paesi: quello con la Francia, per esempio, risale al 1989; quello con il Principato di Monaco è del 2015. Questa può essere l'occasione per avviare un ragionamento più complessivo sulla situazione dei lavoratori frontalieri italiani in tutti i Paesi confinanti. L'auspicio è che il passaggio di oggi, anche con un voto all'unanimità trasversale delle forze politiche, possa aiutarci a affrontare i temi dei lavoratori frontalieri. Questo è il merito della discussione di oggi, al di là delle rivendicazioni di parte, che io capisco ma che in realtà, in questo caso, hanno sinceramente poco senso. Oggi l'atto dovuto è per chi lavora quotidianamente attraversando il confine di territori che devono devono essere sempre più integrati e sempre più oggetto di accordi bilaterali per evitare disparità di trattamento.

Quindi, l'Accordo e il Protocollo di cui parliamo interessano un numero di italiani molto significativo, ai quali va data la giusta attenzione. Si tratta di lavoratori che hanno scelto la strada - è proprio il caso di dirlo - del lavoro oltre confine. Si tratta di lavori che, a parità di mansioni, sono di norma pagati molto meglio che in Italia, anche e non solo per il sistema fiscale più favorevole. Sono remunerati al lordo, in quanto in Svizzera non esiste il sostituto d'imposta. Ed è presente un sistema di tassazione e di previdenza sociale che prevede un meccanismo differente da quello italiano: più responsabilizzante, oltre che più conveniente, anche se sulla tassazione svizzera pesano le imposte federali, quelle cantonali e quelle comunali, ma con un sistema di servizi offerti qualitativamente migliore di quello italiano. Quindi, quella al nostro esame è la ratifica di un Accordo e di un Protocollo siglati due anni fa, i quali vanno a modificare l'intesa attualmente vigente, che risale a quasi cinquanta anni fa. La modifica ora proposta viene affrontata dopo che le norme in essa contenute sono stato oggetto di un confronto tra i tre Cantoni svizzeri interessati, le autorità italiane e l'Associazione dei Comuni italiani che sono a ridosso della frontiera, nonché le organizzazioni sindacali. Si intende eliminare la doppia imposizione sulle imposte prelevate nell'altra Nazione, prevedendo che sia lo Stato in cui il lavoratore risiede ad applicare le proprie imposte sui redditi. È ovviamente previsto anche un periodo transitorio per passare dal regime fiscale vigente alla nuova disciplina, a garanzia dei lavoratori e a tutela dei bilanci dei Comuni di quella fascia a ridosso del confine svizzero che sono interessati dal fenomeno dell'esodo quotidiano dei frontalieri. Il problema dei frontalieri riguarda, oltre la Lombardia, la Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano, anche la mia Regione, il Piemonte, con numerosi lavoratori che, dai Comuni della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, si recano in Svizzera ogni giorno. Il tema, molto sentito in Piemonte, è stato affrontato anche dal Consiglio regionale del Piemonte per quanto riguarda i trattamenti speciali di disoccupazione, perché uno dei temi che anche il provvedimento in esame affronta è quello degli ammortizzatori sociali che devono essere attivati nei confronti dei frontalieri che perdono il lavoro. Sono disposizioni che riguardano tutti i lavoratori. Ma ricordo che va evidenziata una sensibilità particolare verso quei lavoratori che, ultra cinquantenni, si trovano, nei periodi di crisi economica come quella in cui viviamo, senza lavoro e hanno assoluta necessità di vedere applicati nei loro confronti gli ammortizzatori sociali. Ben venga, quindi, che nel provvedimento sia previsto per i frontalieri un'indennità speciale di disoccupazione, che ha lo scopo di attutire gli effetti negativi dei periodi più difficili. Appare però evidente che, nel momento in cui si interviene per risolvere le problematiche affrontate nell'articolato che andiamo ad approvare, bisogna forse considerare anche altri problemi. Ad esempio, così come è stato proposto in alcuni ordini del giorno, è assolutamente necessario implementare i nuovi accordi con la Svizzera per agevolare il ricorso al telelavoro nel modo più ampio possibile. Dobbiamo anche interrogarci su quale sia il modo migliore di tutelare il lavoro e il reddito dei territori di confine, e quindi in che modo introdurre forme di fiscalità agevolata per i territori che si trovano a ridosso di aree che hanno un fisco meno pesante. Sarà, quindi, necessaria in futuri provvedimenti introdurre un'ulteriore e più marcata fiscalità agevolata a favore delle imprese dei Comuni delle vallate a ridosso del confine, in modo che possa costituire un volano allo sviluppo economico delle nostre imprese di quei territori e ridurre la propensione allo spopolamento delle nostre aree montane, creando maggiore occupazione. Le norme del disegno di legge in esame certamente segnano un passo in avanti, evitando la doppia imposizione e introducendo un sistema di tassazione concorrente: un fatto nuovo e importante dopo tanti anni. Ed è per questi motivi che esprimo il convinto voto a favore del Gruppo Forza Italia. Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà a favore della ratifica, ricordando che questo provvedimento arriva da lontano e ha visto impegnati diversi Governi, da ultimo il Governo Conte 2.

pandemia. Come MoVimento 5 Stelle speravamo di arrivare in Aula addirittura senza alcun emendamento e alcun ordine del giorno. Per la prima volta dopo molti anni, ho visto le Commissioni congiunte 3a e 6 a un parere pressoché unanime sul provvedimento; quindi, ci è sembrata abbastanza assurda la quasi polemica del senatore Romeo che ha voluto rivendicare la genesi. Eravamo tutti d'accordo, ci sembrava cosa buona e giusta per i lavoratori; non mettevamo bandierine, nessuno lo ha fatto, per cui a noi è sembrato un po' fuori luogo. Capiamo che in Lombardia ci saranno le elezioni; capiamo che bisogna spingere Fontana; capiamo tutto, ma, forse, non era né il momento né il luogo per fare questo tipo di rivendicazione.

Tenevo però ad evidenziare l'aspetto ambientale che si è determinato con la mancanza di traffico e di spostamenti tra Italia e Svizzera nel periodo della pandemia, potrebbe essere in realtà un bel volano ambientale. Gli ordini del giorno che abbiamo presentato andavano esattamente in quella direzione:

per evitare che si usassero fonti fossili e per procedere a una protezione dell'ambiente molto più spinta, molto più coraggiosa. Questo era ed è un piccolo passo,

e buona è stata quella di attuare un doppio binario, quindi di non penalizzare gli attuali frontalieri finché non andranno in pensione, con un binario diverso per i nuovi. Ne abbiamo discusso con l'ambasciatrice svizzera e con le autorità svizzere,

avvantaggia i lavoratori frontalieri (anche quelli che rimangono a lavorare in Italia) altrimenti ci sarebbe il rischio di svuotamento di una zona cuscinetto. Se me lo consentite, apro una piccola parentesi.

ad attivarsi per far uscire definitivamente la Svizzera dalla *black list* italiana, perché ormai i tempi sono maturi, come ha detto anche il presidente della Repubblica Mattarella. Le autorità svizzere si sono impegnate tantissimo e ci sono tantissime forme di collaborazione, per cui penso che anche questo secondo tassello, oltre alla tassazione dei frontalieri, possa avere a breve una felice conclusione. *(Applausi)*. vorrei partire dal contesto nel quale ci accingiamo ad approvare la ratifica di un accordo fiscale fra Italia e Svizzera atteso da tempo, perché i primi accordi

territorio che vive del rapporto con la Svizzera, in particolare con il Canton Ticino. In quel 1974 fu il sindaco di allora di Lavena Ponte Tresa, Antonio Sanna, che è scomparso proprio questa estate, ad ispirare questi accordi.

Allora le persone che varcavano il confine e andavano a lavorare nel Canton Ticino erano 5.000. Quel numero è via via cresciuto e siamo arrivati, proprio in questi giorni, alla cifra *record* di 90.000 lavoratori che passano il confine delle Province di Verbano-Cusio-Ossola, di Varese, di Como, di Sondrio e di quella parte dell'Alto Adige che confina con la Svizzera. È cambiato il mondo e la Svizzera più volte ci ha posto il tema di regolare diversamente i rapporti dal punto di vista fiscale e non è stato facile farlo in questi anni, perché erano tante le resistenze sul territorio e poco avvertiti quei Governi che hanno tentato di cambiare le regole calando dall'alto dei modelli e non costruendone in un rapporto con le realtà territoriali. Parto da qui, altrimenti non si capirebbe perché poi, alla fine, siamo riusciti a trovare un accordo che ha accontentato tutti. ha ricordato il lavoro che ha fatto quando era Vice Ministro degli affari esteri, perché si era parlato, a un certo punto, di una gradualità nella tassazione anche dei vecchi frontalieri. Mi fa piacere che abbia riconosciuto il lavoro fatto in continuità dal senatore Misiani, quando ha ricoperto l'incarico di vice Ministro dell'economia e delle finanze. In quel caso però - lo dico al collega Garavaglia - c'è stato un punto di svolta, perché non è stato solo il lavoro in continuità che aveva giustamente impostato al MEF, e cioè l'idea che si potesse partire - ed è il primo punto fondamentale nel rapporto con gli svizzeri - ponendo due condizioni. La prima è la clausola di salvaguardia, per per garantire tutti i lavoratori frontalieri che avevano iniziato a lavorare con determinate condizioni, avevano fatto progetti di vita e acceso mutui sulla base di quel tipo di tassazione,

non un euro di più di tasse per i lavoratori frontalieri che già lavoravano, non un euro di meno per i Comuni di frontiera che chiudono i loro bilanci grazie ai ristorni. Nell'accordo del 1974 il principio era proprio di essere messi in condizione di dare servizi di base (gli asili, le strade) ai lavoratori che andavano a lavorare dall'altra parte e pagavano le tasse dall'altra parte, ma non c'era la possibilità la possibilità di fargliele pagare in Italia e di mantenere i servizi. C'era una popolazione che cresceva sempre di più e in quei Comuni rappresentava la maggior parte della forza lavoro, che ci viveva e usufruiva dei servizi, ma non pagava le tasse lì e quindi bisognava trovare Queste sono state le due condizioni per aprire il negoziato con la Stoffel e con le autorità svizzere e arrivare a un accordo fiscale equilibrato. C'era poi la seconda parte, che è stata la vera innovazione che ci inventammo allora con Antonio Misiani, un *memorandum* con il territorio, con le forze sociali e con i sindaci dei Comuni di frontiera. È stata quella la vera chiave di volta rispetto al 2015, quando si cercò di imporre un modello sul territorio non negoziandolo e si misero in campo una serie di condizioni, non solo la clausola di salvaguardia per gli attuali lavoratori frontalieri, ma benefici fiscali per i nuovi lavoratori frontalieri che verranno assunti dal 2024, che, innalzata da 7.500 euro a 10.000 euro la franchigia, avranno un *bonus* fiscale di 2.500 euro, destinato non solo ai lavoratori che vanno in Svizzera, ma esteso anche a tutti i lavoratori

con un aumento della soglia - una battaglia che abbiamo fatto noi come Partito Democratico nella passata legislatura - dal 30 al 50 per cento della possibilità di applicarli sulla spesa corrente. Infatti, come dicevo prima, i bilanci di quei Comuni fanno fatica a chiudersi e c'è bisogno di dare risposte

La vera innovazione all'interno di questo *memorandum* è stata però l'istituzione del fondo di cui abbiamo parlato poco fa per lo sviluppo socioeconomico e infrastrutturale delle fasce di confine, perché qui si riconosce per la prima volta in maniera esplicita la specificità di un territorio che, come dicevo prima, esporta lavoratori e importa consumatori, con un effetto di spiazzamento per le imprese che fanno fatica a trovare manodopera qualificata per i differenziali degli stipendi pagati in Svizzera e nelle province di confine. Con l'aggiustamento dell'emendamento che abbiamo approvato oggi si rende ancora più completo quel fondo, che a regime arriverà a più di 230 milioni e potrà essere concertato con le istituzioni del territorio, in modo tale da spenderlo nell'interesse delle comunità di confine. dei territori, il primo esperimento di federalismo fiscale, perché quei soldi rimarranno ai Comuni delle fasce di confine.

a un amico, avversario politico, con il quale abbiamo condiviso questa battaglia, l'onorevole Matteo Bianchi. Penso che sia sintomo di intelligenza politica riconoscere quando si conducono insieme

gli ordini il giorno che tutti insieme, MoVimento 5 Stelle, Lega e Partito Democratico, abbiamo fatto sul telelavoro, perché appunto cambiano le modalità di lavoro, anche oltre l'emergenza. La politica dev'essere in grado di provare a non subire i processi di cambiamento, ma a guidarli. Spero quindi che il Governo risponda velocemente all'impegno che ha assunto oggi in quest'Aula

completamento proprio a causa della conclusione anticipata della stessa. Vale qui la pena di ribadire che i contenuti delle intese bilaterali sono destinati a riformulare

evitando che i lavoratori che risiedono e lavorano in Paesi diversi siano soggetti a doppia imposizione o trattamenti fiscali iniqui, andando tra l'altro a sottolineare l'importanza di un territorio economicamente così virtuoso. È altrettanto bene ricordare che analoghe criticità possono pertanto individuarsi anche con riferimento ad altri Paesi confinanti, come la Francia, più direttamente interessati al fenomeno, o come il Principato di Monaco, dove il regime fiscale dei lavoratori frontalieri richiederebbe un intervento di aggiornamento volto a tutelare maggiormente gli interessi fiscali dei lavoratori coinvolti. Sarebbe pertanto auspicabile che misure analoghe a quelle in esame venissero adottate in tempi brevissimi anche a favore di questi lavoratori frontalieri, ovvero in tutti i Paesi in cui si riscontrano le medesime condizioni oggettive, proprio al fine di rimediare a questa situazione di disparità. Oltre a questo quadro giuridico, che come è stato ribadito elimina le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri, mi preme però sottolineare che proprio in un'ottica di semplificazione, che tutti continuiamo ad auspicare, e di trasparenza, viene introdotto il principio di cooperazione amministrativa, che attraverso le previsioni di uno scambio di informazioni, quali i dati identificativi del lavoratore, i dati sull'ammontare del salario e dei contributi sociali obbligatori, nonché tutti i dati identificativi del lavoratore, consentirà allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero, mediante un flusso elettronico, proprio verso la direttrice della digitalizzazione, di applicare la propria tassazione. modo mi piace sottolineare che assume particolare rilievo l'introduzione di un'apposita disposizione, volta a prevedere la deducibilità dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria, proprio in base a disposizioni contrattuali, che sono a carico dei lavoratori frontalieri. In base a tale previsione, i lavoratori potranno finalmente fruire della deducibilità dei contributi medesimi. Cruciale Grazie,

sull'esperienza intrapresa durante l'emergenza da Covid-19, che ha permesso di sviluppare modalità di telelavoro e, più in generale, di *smart working* moderne ed efficaci, apprezzate da lavoratori e imprese. Tali modalità lavorative hanno generato indubbi vantaggi per la qualità della vita dei frontalieri, unitamente però a sensibili miglioramenti in tema di traffico veicolare e di inquinamento ambientale nelle zone di frontiera

di raggiungere a breve un'intesa positiva, in base alla quale i lavoratori frontalieri possano effettuare la loro prestazione in regime non solo di telelavoro, ma anche di *smart working*, fino a un massimo del 40 per cento dell'orario di lavoro. Tale previsione avrebbe quindi un duplice effetto positivo: portare un beneficio diretto sulla qualità della vita dei lavoratori, il famoso *welfare* sociale di cui sempre parliamo; in secondo luogo, migliorare l'impatto ambientale complessivo, in linea con la nostra convinzione che scelte intelligenti possano dare vantaggi sia alla persona sia al contesto ambientale ed economico di riferimento.

degli organi di stampa, che richiedono risposte chiare da parte del ministro Nordio, non solo quanto alla situazione dell'articolo 41-*bis*, ma anche quanto alla diffusione di una serie di

con un'informativa del Ministro della giustizia sul caso Cospito alle ore 18. I Gruppi potranno intervenire per dieci minuti. Anticipo

piccole modifiche, la prima delle quali, rispetto al finanziamento che era stato pensato per il funzionamento della Commissione, prende atto che l'anno 2022 è già passato, per cui si elimina il finanziamento per il 2022 e si mantiene a 100.000 euro quello per ciascun anno di lavoro. Si aumentano i componenti, dai 16 inizialmente previsti a 18, con la garanzia che ciascun Gruppo, tanto per la Camera dei deputati quanto per il Senato, sarà sempre rappresentato.

Visto che però abbiamo a cuore l'approvazione del disegno di legge in esame nei tempi più brevi possibili, pensiamo che, tutto sommato, non cambiando il senso del disegno di legge, possiamo comunque licenziarlo

Signor Presidente, mi associo alle considerazioni e alle valutazioni della relatrice Valente, che condivido in pieno.

molto atteso. Istituire nuovamente la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere è infatti un importante passo, in questa legislatura, verso obiettivi di giustizia nei confronti delle donne, che dobbiamo perseguire e che non ammettono divisioni. Essi vanno perseguiti con unità di intenti, in continuità con il compito intrapreso dalla precedente Commissione. quindi l'occasione per ringraziare non solo i relatori, oggi, ma anche chi nella scorsa legislatura ha svolto un lavoro importante, per portare alla luce, sulla base di dati verificabili, i problemi e gli ostacoli che ancora oggi, nonostante un buon sistema normativo, le donne che decidono di sottrarsi alla violenza maschile devono affrontare e che a volte, purtroppo, come si sa, portano a esiti tragici. Per superare questi ostacoli, il legislatore deve prima di tutto conoscerli, capire quale impatto hanno sulla realtà vissuta dalle donne e come, nella concreta applicazione delle leggi, ci possano essere smagliature e percorsi che si dimostrano inadeguati. Sappiamo per esempio quanto i pregiudizi culturali siano ancora diffusi anche in sede giudiziaria e inducano troppo spesso a non riconoscere la violenza e a confonderla con un banale conflitto nella coppia, non cogliendo il punto fondamentale, cioè lo squilibrio di potere, che produce violenza e che è anche prodotto dalla violenza, innescando un circolo vizioso. Questo approccio, frutto di incrostazioni culturali diffuse, porta a sottovalutare la violenza, domestica e non solo, e spesso a non credere alle donne, esponendole alla vittimizzazione secondaria, invece di assicurare loro la necessaria protezione da parte delle istituzioni. Tutto questo rischia di scoraggiare le denunce e l'emersione dei fenomeni di violenza, che sappiamo ancora non emergere completamente, con il rischio di ricacciare le donne nel silenzio e persino nella colpevolizzazione. Continua, quindi, ad essere necessario monitorare l'attuazione della Convenzione di Istanbul, perché l'introduzione di nuove fattispecie e l'inasprimento delle pene è fondamentale, ma - come purtroppo dimostrano i numeri dei femminicidi, anche in questa prima parte dell'anno - è un deterrente che va affiancato da altri interventi: per esempio, da un'attenta formazione di tutti gli operatori e il personale coinvolto, dalla magistratura agli assistenti sociali e al CTU. Va individuata e proposta una formazione di qualità che eviti costrutti antiscientifici, cioè non confermati da un percorso diagnostico definito e condiviso dall'intera comunità scientifica. Dobbiamo formare persone che sappiano costruire intorno alle vittime un'accoglienza e un ascolto adeguati. Più volte è stato segnalato anche il rischio della vittimizzazione secondaria, quando si tratta dell'affidamento dei figli minori, richiamando l'applicazione della già citata Convenzione di Istanbul. Abbiamo assistito a provvedimenti che disponevano l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, anche in presenza di madri vittime di violenza. La sottovalutazione dei fatti e del rischio che corrono non solo le donne, ma i minori coinvolti è probabilmente dovuta anche in questi casi a una resistenza di vecchi stereotipi e spesso al mancato ascolto diretto dei minori. Pensiamo sia necessario indagare più a fondo sulle ricadute di queste scelte sui minori e in particolare su quelli trasferiti nelle case famiglia, attraverso una valutazione delle conseguenze e degli effetti degli allontanamenti: un *follow up* sostanzialmente per individuare quali effettivamente siano le buone prassi da seguire. Il Governo da parte sua ha implementato le risorse per i centri antiviolenza già nella recente legge di bilancio.

per affrontare i nodi, le incongruenze e le smagliature ancora presenti nella nostra legislazione. Quindi, sarà oggetto di particolare attenzione da parte del Ministero per le pari opportunità: la presenza, anche indiretta, di forme di mediazione fra vittima e violento; il problema del declassamento della violenza a conflittualità; l'introduzione della valutazione del rischio, lavorando sugli indicatori di rischio, fondamentale per la prevenzione; la violenza assistita e la protezione dei minori; la verifica dei percorsi per maltrattanti con *follow up* che includa la valutazione del pericolo di recidive. È indispensabile riconoscere la dimensione sistemica del fenomeno della violenza contro le donne e mettere in campo un impegno istituzionale di lungo periodo per contrastarla, attraverso un grande cambiamento culturale. Per fare questo serve una campagna forte e unitaria, allo scopo di sradicare la cultura del dominio di un sesso sull'altro e garantire alle donne giustizia e sicurezza. È in quest'ottica di sinergie e di unità di intenti che apprezzo particolarmente l'istituzione di questa Commissione, a cui auguro buon lavoro già adesso

Signora Presidente, colleghi senatori, Ministro, ci risiamo con il macabro *countdown*: Giulia, Martina, Teresa, Yana, Oriana, Giuseppina, sono i nomi delle donne che, solo nel mese di gennaio appena concluso, sono rimaste vittime della follia omicida. Solo qualche mese fa la nostra Assemblea ha votato all'unanimità il rinnovo dell'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio... *(Brusio)*. PRESIDENTE. Mi perdoni, senatrice Biancofiore. Colleghi, ovviamente l'argomento è importante e do per scontato che sia di grande interesse per tutti. Quindi vi chiedo di abbassare molto il volume della voce e di consentire a noi di seguire i lavori e alla senatrice Biancofiore di svolgere il suo intervento.

Come avevo già detto in sede di dibattito sull'istituzione della Commissione, la necessità della reiterata istituzione della Commissione d'inchiesta conferma a tutti noi che purtroppo, nonostante si siano colmati colpevoli ritardi, la cronaca quotidiana ci restituisce una fotografia che parla ancora di fallimento degli sforzi, delle leggi e degli strumenti messi in campo. Questo dato è stato confermato anche in questo inizio del 2023; bisognerebbe fare anche uno sforzo di fantasia. Ho sempre sostenuto che, su un tema delicato come quello del femminicidio, debba essere garantita la massima partecipazione e il coinvolgimento della società civile, che non può che partire dai Gruppi presenti in questa sede. Oggi non posso quindi che salutare con favore la scelta di ampliare la composizione della Commissione, in modo da consentire la partecipazione di tutti i Gruppi parlamentari, compresi i più piccoli come il nostro. La prospettiva e il dibattito su questa tematica devono essere infatti il più possibile inclusivi. Per questo auspico altresì che i lavori che terrà la Commissione consentano la partecipazione, nelle forme più opportune, di tutte le componenti della società, che sia con idee, audizioni di esperti o iniziative specifiche volte alla prevenzione. Il femminicidio non è un argomento da donne o da salotto; è un tumore che coinvolge tutta la società. Garantire la partecipazione ampia anche degli uomini, che sono padri, fratelli e mariti, con molta probabilità potrebbe rappresentare un supporto fondamentale nell'attività di prevenzione. L'intento che ha portato all'istituzione di questa Commissione non è quello di schierarsi a favore o contro un genere, ma proprio quello di studiare il fenomeno e promuovere delle misure incisive che siano il più possibile condivise e che possano fungere da tutela per le vittime. Le cifre delle vittime, che, nella freddezza dei numeri, ci impediscono di provare la stessa empatia che proviamo quando ci confrontiamo con le loro storie, sono spaventose: un omicidio ogni tre giorni. Lo voglio ripetere a tutti: un omicidio ogni tre giorni. Il 2022 non si è chiuso meglio del 2021: dall'inizio di gennaio a fine dicembre scorso sono state oltre 120 le donne uccise; di queste tante, tantissime, sempre troppe, sono vittime degli ex *partner*. I dati resi noti dal Viminale sono agghiaccianti, confrontando i primi mesi del 2022 con quelli del 2021, sebbene si sia assistito ad una diminuzione del 10,3 per cento degli atti persecutori o *stalking* e del 3,9 per cento dei maltrattamenti in famiglia, mentre c'è stato un aumento di ben 15,7 punti percentuali delle violenze sessuali. Questa è la dimostrazione più lampante che quanto fatto finora dalle istituzioni, ma anche, bisogna dirlo, dal contesto sociale, non è sufficiente. C'è il dovere di fare di più. La strada maestra deve essere quella del coinvolgimento: coinvolgere per studiare, coinvolgere per informare, coinvolgere per prevenire, coinvolgere per agire. Oggi, quindi facciamo un altro passo nella giusta direzione, incrementando la partecipazione in ottica inclusiva, perché il tema della violenza sulle donne necessita di un impegno quotidiano, sentito e appassionato, ma soprattutto trasversale, che sappia condizionare il dibattito pubblico, sempre senza distinzione di colore politico, lavorando costantemente

necessità di fare un Consiglio superiore di sicurezza. In tali organi l'interesse di parte non dovrebbe prevalere sull'interesse comune, garantito proprio a partire dalla partecipazione di tutti i Gruppi parlamentari. Agire su queste tematiche cruciali insieme, con il supporto e la rappresentanza di tutti, è un servizio che viene reso prima di tutto al Paese. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati-MAIE al disegno di legge presentato.

una parola che utilizziamo da molti anni, che abbiamo scritto spesso per denunciare quello che accade anche nel nostro Paese, per informare e far capire che quello che avviene attorno a noi spesso non è un caso, non è il frutto di un *raptus* di follia, non è passione, non è gelosia, non è amore. Ma questo sembra non essere sufficientemente chiaro per tanti: per la società civile, per i media e anche per la politica. Noi sappiamo bene che alcune parole spiazzano e a volte fanno anche paura, per la consapevolezza che evocano, per le responsabilità che denunciano. Il termine femminicidio nacque per indicare gli omicidi delle donne in quanto donne. Noi, però, non stiamo parlando soltanto degli omicidi di donne commessi da parte di *partner* o ex *partner*, ma anche, per esempio, delle ragazze uccise dai padri perché rifiutano un matrimonio che viene loro imposto oppure perché rifiutano il controllo ossessivo delle loro vite o delle loro scelte sessuali. In questa scia di crimini, credo che vada detto in quest'Aula che vanno annoverate anche le donne uccise dall'AIDS contratto da *partner* sieropositivi, che per anni hanno intrattenuto con loro rapporti non protetti, tacendo della loro sieropositività; o anche le prostitute contagiate dall'AIDS oppure ammazzate dai clienti, le giovani donne uccise perché lesbiche oppure, come era una volta, tanto tempo fa fortunatamente, le streghe che venivano bruciate sul rogo. Purtroppo, se muore una ragazza di vent'anni, buona ed amata da tutti, merita lo *status* di vittima. Se, invece, muore una prostituta uccisa da qualcuno, forse se lo merita un po' meno. Anche per questo, però, si alimenta il meccanismo della violenza. Sostenere l'idea che, se fossero tutte sante, non correrebbero dei rischi, vuol dire proprio dichiarare l'esistenza di una colpa che giustifica l'atto violento. Lo sanno, peraltro, talmente bene gli uomini che questo è uno strumento potente, che agiscono in maniera sistematica nel percorso violento, alle volte fino al gesto finale. L'antropologa messicana Marcela Lagarde sostiene che con la parola femminicidio si indica un problema strutturale che va al di là degli omicidi delle donne, riguardando, cioè, tutte le forme di discriminazione e di violenza di genere che hanno la forza brutale di annullare la donna nella propria identità e nella propria libertà, non soltanto fisicamente, ma anche nella dimensione psicologica, nella socialità, nella partecipazione alla vita pubblica. È per questo che a mio avviso non basta semplicemente istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio - cosa ovviamente buona e giusta - o appellarsi ai doveri delle istituzioni e dei poteri pubblici, ma occorre qualcosa in più da parte della politica, della cultura, della società in tutti i suoi ambiti, e naturalmente occorre qualcosa in più anche da parte della scuola. Con la legge del 27 giugno 2013 l'Italia ha proceduto, come sappiamo, alla ratifica della Convenzione di Istanbul - il Parlamento all'epoca la votò all'unanimità - che chiedeva agli Stati impegni concreti, tra cui il sostegno e il potenziamento dei centri antiviolenza e un'opera di prevenzione da fare proprio nelle scuole. scuole. Peraltro, tutti coloro che si sono occupati di violenza maschile sulle donne sanno perfettamente come il fenomeno abbia radici culturali profonde e che per poter intervenire in maniera efficace è fondamentale lavorare proprio sulle giovani generazioni, sui bambini, sui ragazzi, su coloro che evidentemente ancora hanno la possibilità di non sedimentare quei pregiudizi e quegli stereotipi di genere che portano guasti indelebili nelle relazioni interpersonali. È esattamente la ragione per cui la Convenzione di Istanbul prevede l'introduzione di una forma di educazione all'affettività nelle scuole, che peraltro è una scelta già prevista dagli ordinamenti di tutta Europa, tranne, però, purtroppo, l'Italia e la Grecia. Sarebbe importante, invece, che l'educazione di genere, l'educazione alla differenza, alla vita emotiva, entrasse a pieno titolo nei *curricula* scolastici, magari non come ulteriore disciplina aggiuntiva, ma come sfondo integrante di tutti i saperi che vengono insegnati e che diventano evidentemente propedeutici ad altri saperi, e anche e soprattutto alla vita. Eppure, da anni, i centri antiviolenza aspettano il finanziamento del Piano nazionale; stiamo parlando, peraltro, di piccole cifre che non sempre arrivano a destinazione. Nonostante qualche timido avanzamento legislativo, dobbiamo sapere che ogni anno si annoverano tra le 100 e le 200 donne che perdono la vita per mano di un uomo. Oggi sicuramente è cresciuta l'attenzione mediatica, ma occorre potenziare la cultura dell'ascolto della vittima, a partire, per esempio, dal riconoscimento che il femminicidio, lo *stalking*, i maltrattamenti, oltre alla violenza sessuale, sono anch'essi forme di violenza di genere rivolti contro le donne in quanto donne, e occorre partire da questo per raccogliere i dati secondo un'ottica di genere, per capire se davvero le donne che chiedono aiuto vengano effettivamente protette o se, invece, vengono lasciate sole, come spesso accade a tutte quelle donne che svolgono lavori precari o mal pagati. Spesso, infatti, come sappiamo, mancano anche i posti letto per accoglierle perché i fondi sono insufficienti e le case di rifugio spesso chiudono. Succede anche che le leggi esistenti vengano male applicate oppure, per esempio, che una donna ricada in una condizione di vittima e che il caso non venga adeguatamente valutato e può succedere per tanti motivi: per esempio, la mancanza di fondi che possano garantire una formazione specifica agli operatori professionali. Succede anche però - è bene saperlo che si verifichino pericolosi ritorni al passato come, per esempio, si legge in qualche disegno di legge di qualche esponente politico della maggioranza (avremo di che discutere). Istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio quindi importante, fondamentale, ma bisogna trovare la strada per svelare efficacemente tutti gli aspetti del problema, richiamare alla propria responsabilità soprattutto gli uomini, quelli che hanno ruoli pubblici, ricoprono cariche di prestigio, che occupano posti di eccellenza. Seppure i passi in avanti in tutti questi anni ci sono stati su alcuni aspetti - per fortuna! - l'attenzione alla formazione e alla protezione delle donne che decidono di uscire da situazioni di violenza deve essere, invece, ancora profondamente tutelata e deve essere evidentemente ancora maggiore. Ancora oggi troppe donne vengono ammazzate perché manca una reazione collettiva a una cultura che spesso è da definire solo come assassina, che riporta in auge pregiudizi e stereotipi antichissimi, legati alla malintesa virilità, all'onore, al ruolo degli uomini e delle donne nella coppia, nelle società. insomma, di questioni che ben conosciamo e che purtroppo hanno a che fare profondamente anche con la storia del nostro Paese. Se oggi le Nazioni Unite parlano di femminicidio è perché in Italia, in Europa, nel mondo, in tantissimi Paesi ci sono state fortunatamente donne che hanno reclamato il riconoscimento, per le donne in quanto donne, di quei diritti umani affermati a livello universale, in particolare del diritto inalienabile alla vita e alla integrità psicofisica. I diritti, però, vivono soltanto laddove vengono reclamati in quanto tali, altrimenti rimangono destinati al mero riconoscimento formale. Per l'Italia credo che questa sia una battaglia di civiltà che riguarda le donne, ma anche gli uomini, la società civile, la politica e le istituzioni ed è per questo che annuncio il voto favorevole delle senatrici e dei senatori della componente dell'Alleanza Verdi-Sinistra. Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, la Commissione parlamentare d'inchiesta che ci accingiamo a istituire si prefigge come prima finalità quella di svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna fondata sul genere e, e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne. Ritengo che il primo e più importante obiettivo da raggiungere sia capire cos'è il femminicidio. Non mi riferisco ovviamente al fatto materiale in sé, all'uccisione della donna, ma a quell'insieme di fattori causali e condizioni sociali, culturali ed economiche a causa delle quali le donne vengono molestate, mortificate, percosse, umiliate, violentate e infine anche uccise. uccise. Il femminicidio, infatti, è l'acme di una serie di atti e condotte che spesso sono protratti per anni o che, in altri casi non meno drammatici, si concentrano nel breve volgere di pochi mesi. che si tratti di una storia di violenze domestiche perpetrate in vent'anni di convivenze o di un rapporto patologico durato pochi mesi, il risultato spesso non cambia: è l'uccisione della donna per mano dell'uomo. Illuminanti sul cammino che questa Commissione è chiamata svolgere sono le conclusioni formulate dalla Commissione del Senato nella passata legislatura, dalle quali emergono due dati sconfortanti: il primo è che il 63 per cento delle donne non aveva mai riferito a nessuna autorità pubblica e neppure a un familiare o a un amico le violenze subite dall'uomo. Il secondo dato è ancora più inquietante e ci dice che il 15 per cento delle donne uccise aveva in precedenza denunciato per altre violenze quello che poi è divenuto il suo assassino. Questi due dati ci dicono allora che bisogna prestare maggiore attenzione alle misure di formazione, di assistenza e di prevenzione. Occorre cioè formare le Forze dell'ordine e gli operatori sanitari, affinché siano in grado di riconoscere i segni della violenza e bisogna evitare che si inneschi l'odioso fenomeno della vittimizzazione secondaria, che si manifesta tutte tutte le volte in cui si chiede alla vittima che cosa abbia fatto per scatenare l'aggressione o, ancora peggio, perché non abbia denunciato prima. Ben vengano allora gli ulteriori obiettivi del disegno di legge, che prevedono che la Commissione indaghi ed accerti anche le possibili incongruità e carenze della normativa vigente per tutelare le vittime della violenza e che indaghi anche per accertare il livello di formazione e di attenzione, nonché la capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni competenti a svolgere assistenza e prevenzione. Sono obiettivi concreti che indagheranno questa emergenza sociale, questo scandalo del XXI secolo in modo pratico, senza teorizzazioni e speculazioni che sarebbero tardive quanto inutili. Certamente l'introduzione della procedura del cosiddetto codice rosso e altri interventi normativi hanno costituito un decisivo passo in avanti, ma, come è noto a tutti, si tratta ancora di procedure che non trovavano un'applicazione adeguata alla realtà del fenomeno del femminicidio e della violenza di genere. poche sono le forze in campo contro un fenomeno che ha assunto la dimensione di un'emergenza sociale diffusa e trasversale, che riguarda purtroppo ogni fascia sociale e ogni fascia di età. Ma se la tutela giudiziaria è stata dotata di strumenti che possono comunque essere perfezionati e rafforzati, ci sono altri due campi sui quali è necessario lavorare da subito: quello economico e quello culturale. I dati ci confermano che in Italia l'occupazione femminile è la più bassa d'Europa e c'è un alto numero di casalinghe senza alcun tipo di tutela economica. Fin troppo spesso la donna vittima di violenza non denuncia perché non ha i mezzi economici per costruirsi un'altra vita o perché addirittura non dispone neanche delle risorse necessarie per acquistarsi un biglietto del treno e scappare via. Questo tema dovrà essere attentamente indagato fornendo risposte che siano da viatico per la nostra funzione di legislatori e contribuiscano a trovare strumenti efficaci e di rapida attuazione per affrancare le donne dalla violenza di genere e impedire che questa poi sfoci in femminicidio. ultimo, ma non per importanza, occorre agire sull'elemento culturale per eliminare ogni forma di disuguaglianza di genere, ogni superfetazione mentale a causa della quale ancora oggi la donna viene percepita come oggetto di dominio o di desiderio sessuale. Vi è una grande responsabilità in ciò anche da parte degli organi di informazione e dei mezzi di comunicazione di massa, dove la donna è spesso ridimensionata a una figura ancillare oppure, ancora peggio, a una dimensione esclusivamente corporea nella quale conta solo l'apparenza, che a sua volta incoraggia a pensare che vi sia sempre una disponibilità da parte di quest'ultima ad assecondare la volontà dell'uomo. Per non parlare poi di ciò che circola su Internet e sui *social media*, dove giornalmente si scatenano campagne denigratorie e di istigazione all'odio e alla violenza contro la donna, in un clima di sostanziale impunità. Uno dei punti centrali del lavoro che sarà chiamata a svolgere la Commissione riguarda il riconoscimento di alcune forme specifiche di violenza *on-line* come la diffusione di materiale intimo e privato avvenuta in modo non consensuale, il *cyberstalking*, le molestie informatiche e l'incitamento all'odio e alla violenza in Rete. Vanno quindi estesi i reati connessi all'odio e all'incitamento all'odio razziale anche rispetto alle donne, per rafforzare l'intero quadro giuridico della tutela contro ogni forma di violenza di genere. Nel mondo, Presidente, da tempo immemore guerre e conflitti si combattono sul corpo delle donne. Le immagini e le informazioni che ci arrivano dagli scenari di guerra ci raccontano quanta sofferenza subiscano le donne da parte del regime talebano, che le priva della loro dimensione pubblica, relegandole a una dimensione privata in cui sono prive di ogni diritto. E che dire della guerra in Ucraina, combattuta sul corpo vilipeso e violentato delle donne ucraine da parte di un esercito che usa lo stupro come strumento di guerra? E della feroce repressione iraniana che si accanisce sul corpo delle donne che subiscono atroci torture e violenze? Molto concretamente dobbiamo operare affinché tutti i Paesi europei e la stessa Commissione europea ratifichino la Convenzione di Istanbul. Non a caso, ciò costituisce il secondo obiettivo di questa istituenda Commissione parlamentare. Non si si tratta quindi di un tema secondario, ma appartiene alla credibilità di un'Europa come faro nel mondo del rispetto dei diritti universali. Allo stesso tempo, bisogna aggiungere la violenza contro le donne all'elenco dei reati di dimensione europea sancito dai Trattati, in modo che tali reati non restino impuntiti in nessuno degli Stati membri. Per concludere, Presidente, naturalmente il Gruppo per le Autonomie esprime un voto di convinta adesione all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, con una piena e consapevole condivisione degli obiettivi che la Commissione intende perseguire e che guideranno e orienteranno le scelte che poi verranno fatte dal Parlamento e dal Governo

Signor Presidente, con il voto di oggi diamo definitivamente il via alla costituzione della Commissione di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere. Martina Scialdone, Vanessa Zappalà, Caterina D'Andrea, Alessandra Matteuzzi, Anastasia Alashri e potrei purtroppo continuare. Facciamo i conti ogni giorno con storie drammatiche che ci impongono di agire e di farlo in fretta e anche in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario il presidente della Corte di cassazione Pietro Curzio ci ha ricordato quanto sia urgente intervenire su questa materia. Lo ha fatto con un dato che ci deve far riflettere, perché mentre gli omicidi volontari si sono nel tempo progressivamente ridotti, resta invece un'ombra inquietante (così l'ha definita il primo Presidente della Corte di cassazione): circa la metà degli omicidi dell'ultimo anno sono avvenuti nell'ambito dei rapporti familiari ed affettivi e una parte molto consistente - 122 su 310 - vede come prima vittima una donna spesso ad opera del *partner* o dell'ex *partner*. Il dato è ormai costante, anche se proprio nell'anno appena concluso in leggera flessione. purtroppo credo che dobbiamo riflettere, oltre ad avere la consapevolezza che la minaccia della sanzione penale non è evidentemente un deterrente sufficiente a fermare questo orribile fenomeno. È proprio questo che ci indica la strada da percorrere, che non è solo quella penale. Occorre - lo diciamo sempre - una svolta culturale; lo abbiamo ribadito anche nel corso del dibattito su questo provvedimento in prima lettura e lo ripetiamo oggi, perché questa è la ragione che ci spinge ad analizzare il fenomeno e a cercare risposte ulteriori ulteriori oltre a quelle che abbiamo provato a dare in tutti questi anni. Del resto non c'è solo il fenomeno orribile del femminicidio; c'è la violenza di genere quotidiana, che si manifesta sotto molte forme. Ogni giorno 86 donne sono vittime di violenza di genere. Gli autori sono spesso facilmente rintracciabili e questo rende ancora più odioso questo fenomeno, perché gli autori sono gli uomini che hanno spesso un legame sentimentale con queste donne: un compagno, un marito, un ex compagno, un ex marito; alcune volte si tratta di pretendenti rifiutati, sempre persone in qualche modo note alle vittime e alle loro famiglie, il più delle volte persone facilmente identificabili. Nella precedente legislatura, com'è noto, il solo Senato aveva deliberato l'istituzione di una Commissione

di aver dato documentazione utile per poter affrontare e combattere i femminicidi e la violenza di genere. *(Applausi)*. Quella Commissione ha indagato sull'impatto delle misure di contenimento sanitario del Covid sulle violenze domestiche, sul finanziamento e la *governance* dei centri antiviolenza e su questo voglio spendere una parola. Servono finanziamenti strutturali. Troppe volte lo Stato non riesce a combattere i femminicidi centri antiviolenza che vengono finanziati privatamente, purtroppo senza risorse strutturali e non sempre quei volontari sono in grado di aiutare tutte le donne che hanno bisogno. quella Commissione ci responsabilizza, mettendo a disposizione un patrimonio di informazioni, di dati e di analisi che però non esaurisce e non può esaurire l'azione di contrasto a un fenomeno che è ben lungi dall'essere sconfitto. Voglio ricordare un lavoro trasversale che è stato fatto nella legislatura. Mi riferisco all'approvazione del codice rosso, che ha rafforzato le tutele delle vittime di reati violenti di natura sessuale e domestica e ha introdotto alcuni nuovi reati: il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (mi riferisco al *revenge porn*) al *revenge porn*) e il reato di costrizione al matrimonio. Si tratta di un apparato normativo apparentemente imponente, con anche un aumento delle pene per i reati più frequentemente commessi, che però non ha del tutto risolto il problema della violenza di genere.

del lavoro che andremo a fare, grazie anche a un provvedimento che è stato proposto dalla presidente della 2a Commissione, la collega Bongiorno, che prova a introdurre alcune modifiche che vanno nella direzione di rafforzare e di rendere effettivo il codice rosso. Su questo punto ci siamo, anche se siamo all'opposizione e riteniamo che alcune modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale, in materia di avocazione delle indagini, possano essere utili per rendere effettive le misure del codice rosso. Ci auguriamo inoltre che quella sia l'occasione per confrontarsi rispetto ad altri testi che non sono stati approvati nella precedente legislatura: mi riferisco ad un provvedimento che, con tutte le Ministre del Governo Draghi e in particolare con la collega ministra Bonetti, avevamo presentato che è stato approvato in Consiglio dei Ministri. *(Applausi)*. Mi auguro che l'analisi del provvedimento della collega Bongiorno sia anche l'occasione per condividere quel testo e per portare avanti alcune misure che vanno nella stessa direzione, ovvero di non piangere le vittime di femminicidio, ma di evitare che ulteriori femminicidi accadano In conclusione, segnalo che la Camera dei deputati ha utilizzato questo veicolo normativo anche per modificare la composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo Commissione possa vedere la luce, perché stiamo per votare in due Regioni, che rappresentano un quarto della popolazione italiana, senza che si sia insediata la nuova Commissione di vigilanza e quindi mi auguro che,

Il nostro sarà nuovamente un voto favorevole, con un appoggio convinto al disegno di legge, alla Commissione e alle ragioni che ne sostengono la nuova istituzione. È di poche ore la notizia che Maria Amatuzzo, ventinove anni, che è stata uccisa con 12 coltellate all'addome dal marito, alla vigilia del Natale 2022, a Marinella di Selinunte, aveva subito un tentativo di strangolamento già nel maggio 2021. Maria aveva puntualmente denunciato il marito, che era andata a trovarla a Partanna, dove era già ospitata in una comunità, insieme alle due figlie, e mentre tentava di strangolarla con una corda il marito le gridava: "Questa è la tua fine!". Quindi le denunce erano state presentate, la protezione era stata attivata, la nuova denuncia di tentato omicidio era stata presentata, ma tutto questo non è bastato a fermare la mano omicida del marito. Ecco perché il lavoro da fare è ancora molto e gli strumenti da mettere in campo per garantire chi attiva un allarme di pericolo di vita devono essere affinati e resi più efficaci. Le precedenti Commissioni, che erano state costituite presso il solo Senato, hanno certamente evidenziato, attraverso il lavoro e le relazioni prodotte, quanto sia importante tenere alta la guardia sul fenomeno del femminicidio. Ora la Commissione diventa bicamerale e quindi potrà avere una rappresentanza parlamentare più ampia e degli spazi di azione più vasti per indagare sui delitti commessi contro le donne e sulle soluzioni per limitarli. Quando si uccide una donna si va oltre l'omicidio, ma si vuole eliminare non solo una figura femminile, una donna, una mamma, ma spesso quello che ella stessa rappresenta, ovvero la continuità della vita, come nel caso di Maria Amatuzzo. Il femminicidio non va quindi considerato un fatto statistico, ma dietro c'è la volontà di annullare una vita, la sua storia, il suo vissuto, la sua famiglia, perché gli omicidi di donne sono quasi sempre commessi dagli uomini: in questo sta la differenza fra omicidio e femminicidio. Il femminicidio è identificato come tale, perché appunto è ad opera di un uomo, il più delle volte commesso da un soggetto che non vuole accettare che una relazione possa finire. Assieme alle donne che sono le vittime, spesso a saldare il prezzo sono i figli delle vittime, quando non solo loro stessi a pagare con la vita. Ma quando rimangono orfani, oltre ad avere perso la madre, perdono anche la figura paterna, che dopo il delitto ovviamente finisce in galera. Gli orfani del femminicidio in Italia sono più di 2.000, storie di minori o di ragazzi la cui vita sarà tormentata dalle scene indelebili che hanno dovuto subire, assieme ai traumi che li accompagneranno per sempre. Ecco che allora non si parte da zero, ma dal lavoro importantissimo svolto anche nella scorsa legislatura dalla Commissione monocamerale del Senato. Il lavoro della Commissione è documentato da decine di audizioni, quindici relazioni, inclusa quella finale, che hanno esplorato l'efficacia delle misure già adottate e delle disposizioni che potrebbero essere messe in atto normativo, compresa l'adozione di un testo unico in materia di violenza di genere. Questo credo debba essere il ruolo più importante della Commissione della XIX legislatura: individuare un complesso di norme che intervengano per limitare il numero di donne ammazzate, misure che possano agire innanzitutto sulla prevenzione e sulla formazione; quindi, misure che possano allargare le possibilità di protezione e di supporto delle donne, perché siamo certi che la sola punizione del femminicida, che avviene solo dopo, non possa essere lo strumento risolutivo. Il lavoro è quello di monitorare l'efficacia delle misure finora adottate, in tanti anni di omicidi di donne, uccise solo per il fatto di essere donne. Va verificata l'adeguatezza di tutti gli strumenti sinora messi in campo a sostegno delle donne, che vanno migliorati proprio sulla base dell'esperienza e alla luce della loro applicazione. Poi, bisogna adottare procedure che proseguano con l'individuazione più puntuale di norme che possano inchiodare alcuni soggetti alle loro responsabilità.

Oggi un femminicidio ogni dieci viene preceduto da una misura di tipo cautelare per vietare l'avvicinamento, per evitare alle donne l'ultimo incontro con il loro assassino. Inoltre, è importante che le procure di tutta Italia siano a conoscenza delle denunce e, soprattutto, che mettano a conoscenza comune i dati sui precedenti procedimenti penali per la violenza di genere. Molto semplicemente, bisogna creare un *database*, dove poter attingere nel momento in cui si adottano provvedimenti giudiziari. Se il tribunale civile e il tribunale dei minori non hanno una condivisione dei dati, può succedere - com'è successo che in casi di separazione, con denuncia di violenza e maltrattamenti della donna, il tribunale dei minori abbia previsto l'affido condiviso. Proteggere la donna spesso significa proteggere soprattutto suo figlio, prima che sia troppo tardi per poterlo fare. Anche se ogni femminicidio è un femminicidio di troppo, siamo consapevoli che oggi non si parte da zero. Il dato dell'ultimo anno mostra fortunatamente, forse anche grazie alle misure finora adottate e a un'accresciuta sensibilità del Paese, che i femminicidi sono meno di quelli dell'anno precedente, seppure sempre ancora troppi. Va ulteriormente potenziato il sistema di protezione delle vittime e la previsione di strumenti che permettano alle donne il reinserimento nel mondo del lavoro per ottenere l'autosufficienza economica. Quindi, va ampliato il novero delle misure di prevenzione; occorre potenziare i centri antiviolenza, le case rifugio e il sostegno psicologico; va implementato il cosiddetto codice rosso, prevedendo la protezione personale nei confronti delle donne che denunciano, nei casi in cui si palesi per loro una minaccia concreta. Soprattutto, va fatto ancora un lavoro enorme di sensibilizzazione nei confronti delle nuove generazioni: un lavoro lento, ma costante che deve partire dall'informazione e dalle scuole.

e le sue due figlie, che hanno perso una madre e non possono più contare su un padre e con lei ricordare tutte le donne sacrificate senza una ragione. Forza Italia, come ha affermato la nostra capogruppo Senatrice Ronzulli in sede di dichiarazione di voto in prima lettura al Senato, è pronta a dare il proprio contributo per vincere una guerra che deve essere combattuta su più fronti, a cominciare dall'impegno delle istituzioni: un impegno che non può e non deve avere appartenenza, né colori politici e di fronte al quale non esistono maggioranza e opposizione. *(Applausi)*. Ne ha facoltà. LOPREIATO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi e colleghe, cos'è il femminicidio? È ogni forma di violenza fisica e psicologica esercitata e perpetrata sulle donne, onde poterle vedere prima assoggettate e poi deciderne la morte. Nel 2022 sono stati ben 120 - ripeto 120 - i casi di femminicidio nel nostro Paese e già 5 dall'inizio del 2023: donne uccise principalmente dai mariti e dai compagni all'interno delle mura domestiche, luogo che per definizione invece dovrebbe essere sicuro. È chiaro ormai che è fondamentale un cambio di rotta rapido e incisivo. Bisogna intervenire in maniera strutturale e trasversale. Il femminicidio è un dramma dalle molteplici facce. Prima di tutto bisogna cambiare e far nascere un nuovo senso comune, iniziando dalle scuole dell'infanzia. Spesso semplici comportamenti di uso quotidiano sono espressione di un retaggio culturale indirizzato ancora a una sottomissione e svalutazione delle donne. Bisogna *in primis* quindi educare i nostri giovani a un nuovo e più giusto senso del rispetto della donna e dell'uguaglianza di ogni individuo. Dietro semplici battute sarcastiche si nascondono le basi per un atteggiamento discriminante. La violenza sulle donne si combatte prima di tutto creando una nuova coscienza. Ricordiamoci che oggi dobbiamo essere protagonisti di una normativa ben lontana da quella pregressa, assolutamente inaccettabile. Ricordiamo per esempio il matrimonio riparatore: gli stupratori potevano evitare la condanna sposando le proprie vittime. E le donne vittime? Una ragazza che si rifiutasse di sposare il proprio stupratore era considerata una poco di buono. Franca Viola, nel 1965, fu la prima a dire "no", a ribellarsi a questo sistema tribale. Dobbiamo attendere il 1981 per vedere abrogata tale norma. Solo nel 1996 lo stupro non sarà più considerato reato contro la morale pubblica, ma contro la persona. Tanto ancora si deve fare. fare. È ora di mettere in atto politiche di rieducazione, anche sugli stessi autori di violenze. Ma vorrei soffermarmi nel farvi riflettere anche sulle violenze psicologiche. Esistono centinaia di casi in Italia di donne abusate psicologicamente, senza violenza fisica; qui per assurdo risulta ancora più difficile intercettarle e sostenerle. Le stesse donne devono spesso prima superare il pregiudizio e l'incredulità di parenti e amici, che magari le definiscono eccessive o, peggio ancora, insofferenti a comportamenti comuni ed equivocabili. Per questo è fondamentale un intervento nelle scuole affinché le giovani donne possano conoscere e riconoscere sin dai primi segni i comportamenti abusanti; solo così potranno tutelarsi dalla possibilità di incorrere in questi eventi. Che possono essere un giorno amici, conoscenti, parenti, persone vicine che conosceranno il fenomeno e sapranno aiutarle nel ricercare il giusto sostegno, così da evitare di incorrere in situazioni che, nella migliore delle ipotesi, lasceranno indelebili ferite nella loro psiche e nella loro capacità di relazione. In poche parole, bisogna creare giovani consapevoli. Non esiste una sola soluzione. Certo, molto si è fatto con l'istituzione del codice rosso, la legge che prevede l'introduzione di una corsia veloce e preferenziale per le denunce e le indagini riguardanti i casi di violenza contro le donne o i minori. Ma spesso, nonostante tutto, i tempi lunghi e il semplice divieto di avvicinamento non evitano il concretizzarsi di tragedie annunciate. Bisogna anticipare al massimo il momento in cui il soggetto maltrattante sia messo in contatto con la pubblica autorità. La condotta di tali soggetti, infatti, prevede un'*escalation* di condotte: si parte da quelle con gradi di offensività minimi, come ad esempio la ridicolizzazione, per poi proseguire con insulti, minacce e percosse, fino ad arrivare a gesti estremi. Bisogna anticipare anticipare l'intervento già quando si è in presenza di reati spia. Per questo occorre dotare l'ordinamento di tutti quegli strumenti anticipatori che consentono di arrestare questa progressione di condotte aggressive. Presentare il soggetto di fronte al questore, affinché si proceda ad ammonirlo rispetto alle condotte poste in essere, può arrestare questa deriva comportamentale, che altrimenti sfocerebbe verso più tristi conclusioni. In più, raccordare talune ipotesi di reato all'applicabilità delle misure di prevenzione amplifica notevolmente i margini di tutela delle vittime di comportamenti devianti, offrendo, anche in questo caso, un'anticipazione di tutela. In tali casi, infatti, la sorveglianza speciale potrebbe essere disposta anche unitamente all'applicazione dei braccialetti. Proprio in relazione a questi ultimi occorrerebbe valutare la possibilità di applicare su larga scala dispositivi di geo localizzazione, oltre ai braccialetti, in modo tale che la vittima conosca sempre l'esatta posizione del soggetto maltrattante, così da attivare prontamente le Forze dell'ordine nei casi di avvicinamento di questi. Tali dispositivi sono largamente utilizzati in Spagna e hanno ridotto drasticamente la violenza nei confronti delle donne. Il diritto alla vita è sicuramente preordinato rispetto alla tutela della *privacy*. Ovviamente, oltre alla prevenzione bisogna intervenire, in maniera strutturale, anche sul contrasto della recidiva, altissima per questo tipo di delitti. Solo attraverso un compiuto percorso di rivalutazione della condotta è possibile azzerare qualsiasi ipotesi di recidiva. Un soggetto non perfettamente riabilitato e rieducato ricade in questo genere di condotte. A tal fine, occorre dare sostegno ai centri antiviolenza. Spesso, i fondi destinati agli stessi sono insufficienti e soprattutto di breve durata, non rendendo così possibile offrire servizi di assistenza costanti e duraturi alle donne vittime di violenza; violenze che spesso durano da decenni e modificano il senso e la percezione, creando ferite molto profonde nella psiche delle donne abusate, che quindi necessitano di un'assistenza più costante e più duratura. Sostegno che va allargato ai bambini che vivono in contesti abusanti e che subiscono violenze psicologiche enormi. Non possono certo bastare poche sedute per aiutare queste donne e i loro bambini ad uscire dalla tragedia vissuta. Altro tema fondamentale è rendere economicamente autonome le donne vittime di violenza.

Sì, perché questi uomini è in termini di preda che vedono le donne. Si rende, quindi, necessario far sì che sempre più le politiche sociali verso le donne dispongano di mezzi economici sufficienti per poter avviare la loro formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro. lavoro. Solo dieci minuti non sono sufficienti a elencare le questioni che necessitano di una immediata attenzione. Attenzione che sarà massima nel corso dei lavori della neocostituita Commissione di inchiesta:

Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, le discriminazioni di genere, gli stereotipi sulle donne radicati nel substrato socio-culturale, la divisione di ruoli e l'esistenza di relazioni di potere disuguali tra donne e uomini sono fattori che costringono la donna a permanere in una condizione di subalternità in cui si alimenta il ciclo della violenza. I femminicidi sono pertanto gesti estremi di questa natura, che sottendono una realtà complessa di oppressione, di disuguaglianze, di abusi, di violenza e di violazione sistematica dei diritti delle donne. I primi riferimenti ufficiali al termine femminicidio si ritrovano all'interno della risoluzione del Parlamento europeo dell'11 ottobre 2007 sugli assassini di donne in Messico e America centrale e sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro questo fenomeno, nonché nel rapporto annuale sui diritti umani rappresentato dal Parlamento europeo nel 2010, in cui se ne ribadisce la condanna. Di femminicidio si discute, poi, nelle linee guida dell'Unione europea sulla violenza contro le donne, adottate dal Consiglio nel 2008, e nel giugno 2010 l'alto rappresentante dell'Unione europea Catherine Ashton, esprimendo le proprie preoccupazioni sui femminicidi in America Latina, ha definito tutte le forme di violenza di genere come aberranti crimini di femminicidio. La prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica sono i principi cardine della Convenzione di Istanbul, firmata l'11 maggio 2011, che ad ora rimane probabilmente uno dei trattati più impattanti a livello mondiale per il rispetto dei diritti umani dal punto di vista giuridico, culturale e politico. Per la prima volta, la violenza contro le donne viene definita come una violazione dei diritti umani, una forma di discriminazione; si stabilisce che lo Stato, che non fa abbastanza per rispondere a situazioni di questo tipo, deve essere ritenuto responsabile di questa violenza. I suoi obiettivi - le famose quattro P - sono: prevenire la violenza, proteggere le vittime, perseguire penalmente i loro aggressori e attuare politiche integrate. esorta e monitora i firmatari affinché adeguino le proprie leggi prevedendo tutte le nuove fattispecie di reato individuate: non solo la violenza fisica, quindi, ma anche psicologica e connessa alle costrizioni sociali. La Convenzione di Istanbul ha come obiettivo quello di rendere intollerabile la violenza di genere, getta le basi per rendere più sicura la vita delle donne all'interno e all'esterno delle mura domestiche e dei confini europei. Il Trattato è stato infatti ratificato da Paesi dell'Unione europea, ma anche extracomunitari, dal momento che il Consiglio d'Europa è un organismo allargato a 47 Stati membri. Allarma il fatto che, per la prima volta, un Paese firmatario come la Turchia decida di sfilarsi. È doveroso, quindi, non dare nulla per acquisito o scontato, ma, anzi, è necessario mantenere sempre alta l'attenzione su quelli che sono fenomeni lontani dall'essere superati. La violenza di genere è una violenza sessuata, fisica, psicologica, economica, normativa, sociale e religiosa, che impedisce alla donna di esercitare appieno i diritti umani di libertà, integrità fisica e morale; nei casi più estremi è una violenza che arriva fino all'annullamento, all'omicidio. Le vittime di questo tipo di violenza scontano il fatto di avere trasgredito al ruolo ideale di donna imposto dalla tradizione: quello della donna obbediente oppure sessualmente disponibile, di essersi prese la libertà di decidere cosa fare della propria vita. La loro autodeterminazione è punita con la morte da coloro che invece dovrebbero essere più vicini: mariti, padri, fratelli. I dati sugli omicidi sono preoccupanti: si parla di 125 vittime nel 2022. E poi spesso c'è il problema dei figli, di quelli che restano: sono bambini che si trovano senza madre e senza padre - che, non di rado, è anche la persona che ha tolto loro la madre - e a volte senza altre figure familiari di riferimento, oltre che con difficoltà economiche. Quasi sempre per loro, insieme al dolore della perdita e al trauma della violenza di cui sono stati testimoni impotenti, si apre una strada tortuosa, costellata di burocrazia, casa famiglia, affidamenti in prova, tentativi più o meno felici di ricostruirsi qualcosa che assomigli a una famiglia, qualcosa che assomigli a una vita normale. Oltre agli omicidi, vi sono tutti gli atti persecutori, le vessazioni, le umiliazioni, che non sempre vengono denunciate o semplicemente confessati dalle donne. Capita spesso che la violenza domestica venga vissuta come una vergogna e quindi da nascondere; la paura di denunciare di non sapere dove andare e come mantenersi. Quindi, troppo spesso, si vive in solitudine il proprio dramma e, quando si decide di chiedere aiuto, può essere troppo tardi. Abbiamo visto, invece, quanto è importante e necessario intervenire tempestivamente, fin dai primi segnali, nell'interesse della vittima, ma anche del maltrattante, che può essere fermato in tempo. È per questo motivo che, poco più di tre anni fa, il Parlamento ha approvato la legge n. 69. Non a caso il provvedimento viene chiamato codice rosso proprio perché, facendo riferimento a come vengono trattate in un pronto soccorso le persone in pericolo di vita, lo stesso principio vale per quanto viene messo in atto proprio per mettere in protezione le donne che decidono di sporgere il Parlamento è chiamato a dare nuovamente un messaggio di unità nella lotta contro il femminicidio e contro ogni violenza di genere. Lo farà attraverso un voto unanime per l'istituzione della Commissione d'inchiesta che dovrà lavorare su questi temi, analizzare le reali dimensioni e cause dei femminicidio e più in generale di ogni forma di violenza di genere, effettuando un monitoraggio circa la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Dovrà lavorare sulla prevenzione, analizzare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e delle amministrazioni pubbliche competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza. alla realizzazione di progetti educativi nelle scuole, al monitoraggio del lavoro svolto dai centri antiviolenza operanti sul territorio, ivi compresi i centri di riabilitazione per uomini maltrattanti; all'effettiva all'effettiva applicazione da parte delle Regioni del piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie. Questa Commissione dovrà capire e mettere in discussione come il nostro Sistema nazionale è pronto a tutelare le donne vittime di violenza. Annunciando il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, concludo dicendo che il femminicidio implica norme coercitive, politiche predatorie e modi di convivenza alienanti che nel loro insieme costituiscono l'oppressione di genere e nella loro realizzazione radicale conducono alla eliminazione materiale e simbolica delle donne e al controllo del resto. Per fare in modo che il femminicidio si compia nonostante venga riconosciuto socialmente, senza perciò provocare l'ira sociale, fosse anche della sola maggioranza delle donne, esso richiede una complicità e un consenso che accetti come validi molteplici principi concatenati tra loro. Interpretare i danni subiti dalle donne come se non fossero tali, distorcerne cause e motivazioni, negarne le conseguenze: tutto ciò avviene per sottrarre la violenza contro le donne alle sanzioni etiche, giuridiche e giudiziali che invece colpiscono altre forme di violenza, per esonerare chi esegue materialmente la violenza e per lasciare le donne senza ragioni, senza parola e senza gli strumenti per rimuovere tale violenza. Nel femminicidio c'è volontà, ci sono decisioni e ci sono responsabilità sociali e individuali. Le parole dell'antropologa Marcela Lagarde nel lontano 1997 sembrano essere purtroppo attuali, in quanto ci indicano che c'è ancora bisogno di un concreto intervento statale che incida profondamente tale realtà criminale e sociale. Ancora oggi assistiamo - ahimè - a sentenze con sconti di pena, attenuanti generiche, alla giustificazione del movente passionale del *raptus.* che il lavoro della Commissione potrà realmente essere un ulteriore mattone verso la costruzione di una società dove vi siano parità di diritti e una coscienza sociale e civica che faccia breccia nella mente dei nostri giovani ed educhi anche gli adulti alla sensibilizzazione di tale rilevante tema. Ogni donna maltrattata, vessata, imprigionata o uccisa è una sconfitta dello Stato. E fin quando ci sarà qualcuno, magari con la responsabilità di essere un modello per i giovani, che si permette di sghignazzare parlando della scomparsa di una ragazzina di quindici anni, noi dobbiamo essere pronti a condannare quel gesto. Approfitto quindi per lanciare un appello: caro Fedez, abbia la dignità di chiedere pubblicamente scusa a Emanuela Orlandi e alla sua famiglia perché hanno già sofferto abbastanza. *(Applausi)*. inizio questo mio intervento in dichiarazione di voto esprimendo una soddisfazione netta, convinta, se possibile con sobrietà appassionata, al voto favorevole che ci accingiamo a esprimere di qui qualche minuto, probabilmente all'unanimità, per l'istituzione di una nuova Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e contro ogni forma di violenza di genere.

che abbiamo registrato oggi, nelle parole di tutti i Gruppi. Lo voglio dire perché credo sinceramente che quattro o cinque anni fa

è stato fatto un lavoro importante, non credo ascrivibile - sarei troppo presuntuosa - solo alla Commissione parlamentare d'inchiesta uscente. Credo, però, che quella Commissione abbia contribuito a costruire un altro un altro alfabeto sulla violenza maschile contro le donne, che io mi ostino convintamente a chiamare così e a non chiamare violenza di genere per tante ragioni che ovviamente possono essere comprese. Abbiamo costruito un sentire comune - lo dico con sincero apprezzamento - che credo possa testimoniare anche l'onestà intellettuale con la quale non solo io, ma l'intero Partito Democratico approccia la questione, con un sincero apprezzamento anche per le parole espresse dalla ministra Roccella. Non sono parole scontate, così come non era scontato il dibattito in quest'Aula. troppo facile parlare della violenza maschile contro le donne facendo ancora solo riferimento a quanto dovrebbe essere indispensabile inasprire le pene e istituire nuove fattispecie di reato, dicendo che siamo stati bravi a fare tanti passi in avanti su questo fronte.

in termini di impostazione e di impianto giuridico. In questo abisso c'è un lavoro costante e certosino fatto sicuramente innanzitutto - lo voglio ricordare in premessa - dai movimenti femminili e femministi che fuori da queste Aule hanno sollecitato spesso la politica e le donne dentro le istituzioni - e oggi penso di poter poter dire le donne di tutte le forze politiche e finalmente gli uomini - a procedere a una chiara assunzione di responsabilità, affermando innanzitutto che la violenza maschile contro le donne non è più un'emergenza. Oggi ho sentito ripetere tante volte in quest'Aula - non si diceva soltanto quattro anni fa che non è un'emergenza, ma è un fenomeno strutturale legato ai modelli sociali della nostra società; che non è un fatto privato, sebbene si consumi nelle mura domestiche nella stragrande maggioranza dei casi. È invece un fatto pubblico, che quindi interroga e inchioda la politica e le istituzioni all'assunzione di responsabilità, e non è un fatto da trattare come un fatto di cronaca, che oggi più nessuno si sognerebbe di dire che si è trattato di un *raptus*, nessuno più si sognerebbe di dire che quell'uomo che ha ucciso ha avuto semplicemente un momento di cedimento.

di quello che succede fuori da quelle aule. Se oggi ancora troppe volte tante donne vengono ammazzate perché su quell'uomo non è stata fatta un'attenta valutazione del rischio e della sua pericolosità sociale, e quindi non gli è stato messo il braccialetto elettronico, non è vero - e questo per fortuna ormai è patrimonio comune - che che non poteva essere messo quel braccialetto elettronico, come pure addirittura qualche magistrato in qualche circostanza ha detto, perché i braccialetti elettronici non sono disponibili. Il tema vero è che ancora troppe volte nelle aule di giustizia le donne non vengono credute, vengono giustificati i comportamenti degli uomini, si fa fatica a credere a un racconto e, quindi, si fa fatica a leggere la realtà esattamente per quello che è. *(Applausi)*. È per questo che sono importanti le parole che abbiamo sentito oggi pronunciare in quest'Aula. Se posso dire, proprio nelle parole di questo dibattito trovo il senso, la profondità e l'utilità della istituzione di una nuova Commissione parlamentare d'inchiesta alla quale abbiamo chiesto convintamente - tutto il Parlamento si esprimerà probabilmente in maniera favorevole in questo senso

più in profondità, perché il tempo è stato tiranno, soprattutto ovviamente vista la fine prematura della legislatura. Alcune relazioni necessitavano di un maggiore approfondimento: penso in modo particolare a come la violenza impatta sul Sistema sanitario e a come può essere di più e meglio in tutte le agenzie e le istituzioni formative.

delle scuole di ogni ordine e grado e delle università vengano svolti corsi che insegnino ciò di cui discutiamo oggi; o comunque insegnino innanzitutto agli uomini e alle donne ad avere rispetto per la differenza e ai ragazzi più giovani e a tutti quelli che saranno gli operatori di domani ad avere un corretto rapporto gestione del sentimento che si prova per un'altra persona, ma molto spesso anche nella gestione della rabbia, delle emozioni e nel modo in cui si costruiscono rapporti sani in termini di relazione. Io dico che queste relazioni, per esempio, avranno bisogno di un ulteriore approfondimento. Così come dico che ve ne sono alcune che andavano indagate di più: penso alle multidiscriminazioni, alla violenza sulle donne anziane, alla violenza sulle donne disabili e sulle donne immigrate. Ci sono quindi aspetti che possono e devono ancora essere indagati.

i numeri e i nomi che non mi sentirete mai fare inchiodano la politica alle sue responsabilità, penso che la politica debba soprattutto passare oggi da una consapevolezza chiara e diffusa, e quindi, dalle parole ai fatti.

quello che ci preoccupa non è l'impegno sul tema della violenza, perché le parole sono condivise. Quello che ci preoccupa è una visione. Se infatti - come ha detto la ministra Roccella - è la sperequazione di potere causa ed effetto del tema della violenza, bisogna fare attenzione al fatto che questa sperequazione di potere fa i conti con scelte strategiche che mirano in qualche modo ad affermare la donna nella società *(Applausi)*: Opzione donna, la valutazione che viene tolta dal contratto degli appalti sull'impatto di genere all'interno delle aziende,

dal tema della violenza maschile contro le donne. Attenzione a pensare di aggredire il tema della violenza facendo forse il salto di qualità nel passaggio dalla repressione alla prevenzione. Ma la prevenzione è un'idea di donna che abbiamo nella società *(Applausi)*, perché solo così aggrediremo la sperequazione di potere esistente tra gli uomini e le donne, minando quindi alla radice il tema della violenza maschile contro le donne. Ecco la sfida vera a cui - secondo me - siamo chiamati. In questo senso mi permetto di proporre di dare centralità alla voce di tutti quei

che non fanno solo accoglienza e protezione delle donne, ma ci raccontano anche come la violenza maschile contro le donne deve essere letta, raccontata e contrastata. Impariamo da chi ogni giorno quelle donne le accoglie: questo significa sicuramente meno retorica, più fatti e più vicinanza effettiva a chi prova a contrastare la violenza, anche fuori da queste Aule. Mostriamo così il volto bello, serio e rigoroso della politica, che sta ascoltare, si sa mettere in discussione e sa fare un salto di qualità.

l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere. Da quel momento un orologio inesorabile ha segnato, oltre al passare del tempo, anche il verificarsi di altri femminicidi e altre violenze, come ci dicono le pagine di cronaca di queste settimane. Non c'è più tempo, non possiamo più aspettare. Dobbiamo iniziare quanto prima ad analizzare in modo capillare tutti questi fenomeni di violenza, nessuno escluso. escluso. Il femminicidio è soltanto la punta dell'*iceberg*, mentre coperti dalla paura e dalla vergogna gli atti persecutori e i maltrattamenti si consumano quotidianamente nel silenzio. È compito delle legislatore occuparsi non soltanto del fenomeno che si manifesta ed emerge, ma anche del fatto sommerso perché, soltanto una volta portate alla luce, le violenze si possono fermare. Occorre quindi squarciare questa cappa che tutto avvolge e tutto copre, quasi che ciò che non si vede non esista. La donna maltrattata tace e sopporta, perché pensa in fondo di meritarsi quel maltrattamento e questo tabù la tiene prigioniera, prima ancora che del suo aguzzino, di se stessa. Bisogna distruggere questo pregiudizio e ciò si può fare attraverso l'educazione. Se è vero che gli uomini vanno educati al rispetto delle donne, è altrettanto vero che le donne vanno educate al rispetto di se stesse. La rivoluzione culturale che sempre auspichiamo, di cui sempre parliamo, si compie a piccoli passi e il primo di questi passi è comprendere che, prima di essere donne e uomini, siamo persone. Se Se partiamo da qui, non ci sarà più spazio per il sopruso e per la sopraffazione, ma si farà spazio alle differenze, alle peculiarità, alle attitudini, che lungi dall'essere annullate devono essere valorizzate, perché sono ricchezza. Credo che dovremmo fare tutti questo lavoro, senza ideologia, perché non è una battaglia ideologica, ma è una battaglia di giustizia e di civiltà. Gruppo Fratelli d'Italia ne siamo convinti ed è per questo che voteremo a favore.

La seduta è sospesa.

n. 1. Ricordo che, per l'approvazione delle modifiche al Regolamento, l'articolo 64, primo comma, della Costituzione e l'articolo 167, comma 5, del Regolamento prescrivono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Presidente, onorevoli colleghi, con la presente proposta di disposizione transitoria si intende far fronte al contingente problema di rappresentatività del Consiglio di Presidenza che, nella sua composizione, non vede rappresentati alcuni Gruppi parlamentari costituiti nella corrente legislatura. La proposta di integrazione del Consiglio di Presidenza risponde, dunque, alle esigenze di ampliare, limitatamente alla XIX legislatura, la rappresentanza in seno ad un organo le cui funzioni sono di preminente importanza per la gestione del buon andamento dei lavori del Senato. A tal fine, la disposizione transitoria che qui si propone prevede che il Consiglio di Presidenza, su richiesta di Gruppi parlamentari non rappresentati, deliberi l'integrazione del Consiglio stesso con ulteriori senatori segretari in misura non superiore a due. Inoltre, in ottemperanza al principio dell'equilibrio numerico tra componenti e Gruppi di maggioranza e di opposizione, si prevede che, qualora per effetto della suddetta delibera tale equilibrio risulti alterato a svantaggio dei Gruppi di maggioranza, debba procedersi alla elezione di un ulteriore segretario, necessariamente appartenente a un Gruppo di maggioranza. In considerazione della natura transitoria della modificazione proposta e della sua finalità strettamente connessa alle esigenze di una compiuta rappresentatività in seno al Consiglio di Presidenza del Senato, nonché della sua ampia condivisione da parte delle diverse forze parlamentari,

la necessità e la volontà di riconoscere spazi importanti di democrazia, in particolar modo alla minoranza. È una ulteriore dimostrazione di collaborazione e di una volontà, da parte della maggioranza e della Presidenza della Giunta, di voler assicurare le prerogative anche alla minoranza, laddove se ne è ravveduta la necessità. Pertanto, anche con soddisfazione e anche con un condiviso condiviso spirito di collaborazione, che ha unito maggioranza e minoranza, l'approvazione della misura del provvedimento all'unanimità è un segnale molto importante per il prosieguo dei lavori e anche per il clima dei lavori stessi, che potrà vedere

Signor Presidente, il provvedimento che andiamo a votare oggi riequilibra il Consiglio di Presidenza e costituisce un elemento di grande partecipazione alle istituzioni anche da parte delle minoranze. Quello che vi auguro come forza politica è che in futuro non ci siano più quelli che vengono considerati i tagli alla politica. Quest'ultima deve funzionare in modo adeguato e con la partecipazione di tutti; non è un orpello far funzionare bene il Consiglio di Presidenza del Senato. Quindi, mi auguro che alla fine della prossima legislatura non si faccia una votazione populista nel ridurre il numero dei partecipanti solo per dimostrare che si sono tagliati i costi della politica. La partecipazione è fondamentale per il buon funzionamento della democrazia, che a sua volta rende tutti migliori: i cittadini che devono decidere e noi, mettendoci nelle condizioni di far funzionare il sistema.

e cioè deve fare in modo che i Gruppi costituiti a inizio legislatura abbiano almeno un rappresentante al Consiglio di Presidenza. Tra l'altro, sarà una modifica limitata alla

rendendo il Consiglio di Presidenza più rappresentativo e in grado di funzionare in modo migliore. Queste sono le ragioni della nostra posizione favorevole. colleghi, poiché per l'approvazione del testo occorre la maggioranza assoluta dei componenti del Senato, prima di procedere alla votazione finale del documento II, n. 1, dispongo, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, l'accertamento del numero

sono ancora in corso alcune Commissioni che stanno lavorando, e questo rende probabilmente più difficile la presenza in Aula. La pregherei

vorrei associarmi alla richiesta della collega Paita, specificando che semmai si tratta non di una verifica del numero legale, ma del numero dei

poiché per l'approvazione del testo occorre la maggioranza assoluta dei componenti del Senato, prima di procedere alla votazione finale del documento II, n. 1, dispongo, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, l'accertamento del numero dei presenti.

onorevole Nordio, che ringrazio per la presenza e per il rapido accoglimento della richiesta di venire a riferire al Senato sul caso Cospito.

informativa è stata concordata oggi anche per essere simmetrica a quella che ho tenuto fino a mezz'ora fa alla Camera dei deputati. La relazione era stata programmata per informare il Parlamento, con i dovuti dati, essenzialmente tecnici e giuridici, della situazione legata al caso Cospito. Poi, in parte, ma solo in parte, soprattutto negli interventi che sono venuti dai colleghi della Camera, si è allargata, ma tengo a precisare che questa informativa era stata programmata perché era giusto e doveroso informare le Camere - e quindi questo onorevolissimo Senato - di una situazione che è abbastanza complessa dal punto di vista giuridico e umano e che ha sollevato tutta una serie di problematiche negli ultimi tempi, per le quali è bene una *reductio ad aequitatem*, cioè un ritorno all'ordine. per il detenuto Cospito proviamo a partire da una situazione che potremmo definire duplice. Da un lato, Cospito è stato condannato, con una pena che è in esecuzione, trent'anni di cumulo di reclusione, che sta scontando in regime di 41-*bis*. Per questa situazione il ministro della giustizia, presidente Cartabia, durante la precedente legislatura, chiese e ottenne l'applicazione dell'articolo 41-*bis*. La legge dispone che in questi casi l'onere della prova di dimostrare che esistono le condizioni per l'applicazione di questo regime estremamente severo

si è giunti a seguito di emergenze istruttorie dalle quali risulta che il detenuto, inserito al vertice dell'associazione con finalità di terrorismo, ha fornito positiva dimostrazione di essere perfettamente in grado di collegarsi con l'esterno, anche in costanza di detenzione intramuraria al regime ordinario, inviando documenti di esortazione alla prosecuzione della lotta armata di matrice anarchico-insurrezionalista. Con l'ordinanza del 1° dicembre 2022, il tribunale di sorveglianza di Roma (quindi la magistratura) ha rigettato il reclamo presentato dal detenuto

Il provvedimento del tribunale di sorveglianza, molto articolato e complesso, ha stabilito che il decreto ministeriale appare essere immune da qualsiasi censura e che quindi le limitazioni imposte appaiono conformi alla legge e idonee al risultato perseguito. Contro questa ordinanza è stato proposto dal difensore del Cospito ricorso per Cassazione. L'udienza era stata fissata in aprile, ma, a seguito di una richiesta di anticipazione dell'udienza per varie ragioni (che riguardano anche la salute del detenuto), l'udienza è stata anticipata al 7 marzo. Questo percorso esula completamente da qualsiasi giudizio e da qualsiasi valutazione o addirittura possibilità di intervento della politica, del Ministero e del Governo, in ossequio al principio che tutti conosciamo dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. In questo settore è sovrana la decisione della Corte suprema di cassazione, tra poco più di un mese, ed eventualmente poi di quanto seguirà. Il secondo aspetto invece della detenzione severa di Cospito riguarda una richiesta che è stata fatta nel gennaio di quest'anno, sempre dal difensore del detenuto, direttamente al Ministro,

quale devolve o devolverebbe al Ministro della giustizia la possibilità di modificare questo regime, seguendo una determinata procedura. Questo secondo aspetto, che è l'unico che ci interessa, perché è l'unico nel quale possa intervenire il Ministro della giustizia (nel primo, ripeto, è sovrana la magistratura), è quello di cui oggi si discute. L'aspetto più controverso di questo articolo di legge riguarda tuttavia l'intervento di altre magistrature nell'ambito di questa procedura. Mi spiego: se è vero che la decisione finale spetta al Ministro, è altrettanto vero che, secondo questa legge, occorre ottenere preventivamente il parere della magistratura, sia della Direzione nazionale antimafia sia del magistrato di sorveglianza e, se del caso, del magistrato di cognizione. Noi abbiamo ricevuto proprio due giorni fa due giorni fa una richiesta ufficiale del procuratore generale della corte d'appello di Torino, che vi leggo in parte

Cospito «attualmente detenuto nella casa di Sassari, nei cui confronti è in atto, per decreto del Ministro della giustizia, la misura di cui all'articolo 41-*bis*»; poi così «Il mio ufficio - questa è la parte importante - da me personalmente rappresentato, sia nella fase esecutiva sia in quella di cognizione, ha in questa fase il duplice ruolo di pubblico ministero per l'esecuzione e di pubblico ministero presso il giudice procedente». Cosa vuol dire? Il procuratore generale di Torino, in questo momento, riveste un duplice ruolo: è il pubblico ministero presso la fase esecutiva dell'espiazione della pena del Cospito e, nello stesso tempo, però, è il pubblico ministero presso il giudice di cognizione, in quanto Cospito ha pendente un procedimento che lo vedeva imputato per il reato di strage, ma di strage secondo l'articolo 477 del codice penale, per il quale era stato condannato a vent'anni di reclusione. In realtà, il procuratore generale, sempre lui, ha fatto ricorso per Cassazione, chiedendo che questa sentenza venisse cassata o comunque venisse chiesto un rinvio, perché secondo lui era configurabile il reato di strage secondo l'articolo 285 del codice penale. So che sto entrando in argomenti molto tecnici, ma questo è quello di cui vi devo informare. Il reato di strage di cui all'articolo 285 è abbastanza strano, per quanto riguarda la dicotomia tra la rubrica e il contenuto della norma, in quanto si tratta di una strage senza vittime.

La Corte di cassazione, dando ragione al procuratore generale della corte d'appello di Torino, ha richiesto un secondo giudizio, perché, secondo la Cassazione, questi reati commessi da Cospito rientravano nella strage di cui all'articolo 285, cioè in quella punita con l'ergastolo. Questo processo, peraltro, è stato sospeso perché il giudice ha ritenuto di rimettere la questione davanti alla Corte costituzionale. Quindi, il pubblico ministero di Torino, in questo momento, è, come dice lui giustamente, giudice della fase esecutiva della pena in cui si trova Cospito e giudice della fase di cognizione derivante dal giudizio di rinvio dopo la sentenza della Corte di cassazione.

Leggo, perché così siamo più tranquilli: «La questione che mi ha determinato a rivolgermi a lei, signor Ministro, riguarda la possibilità o meno che io sia chiamato ad esprimere un parere in ordine a tale richiesta» - cioè alla revoca del 41-*bis* - «che mira alla revoca della misura, peraltro a distanza di poco tempo dal rigetto del reclamo proposto dal difensore dell'imputato e condannato avverso il provvedimento di applicazione da parte del tribunale di sorveglianza di Roma, su parere conforme della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo». Con un'argomentazione molto ricca - che peraltro vi risparmio - il procuratore generale di Torino chiede, quindi, di poter inviare il suo parere nella sua duplice veste di pm dell'esecuzione e della fase cognitiva. Abbiamo ritenuto che questa richiesta fosse fondata proprio sulla base dell'argomentazione del procuratore generale di Torino, che poi è colui che ha seguito tutti i processi di Cospito, quindi, come recita lo stesso, è colui che conosce meglio di tutti la vicenda.

di recente una busta con un proiettile come minaccia, quindi a lui va tutta la nostra solidarietà di politici e di magistrati. Abbiamo risposto *in die*, come si dice, subito, al procuratore generale, accedendo alla sua richiesta, chiedendogli di inviarci nel più breve tempo possibile questo suo parere. Speravamo che lo facesse entro oggi, ancora prima che fosse fissata la seduta pomeridiana davanti a questo onorevolissimo Senato, ma che almeno arrivasse alle Camere; alle Camere; stamattina ha telefonato dicendo che, proprio per la complessità del parere che sta elaborando, non sarebbe arrivato prima di domani. Nel frattempo, abbiamo ricevuto anche il parere della Direzione nazionale antimafia,

Per queste ragioni il Ministro della giustizia, in questo momento, non è in grado e non ha alcuna intenzione di esprimere una decisione, se prima non ha studiato profondamente i pareri che arrivano da queste autorevolissime magistrature. Questo per quanto riguarda la situazione del 41*-bis* di Cospito;

sono state descritte come condizioni di salute psicofisica discrete e stazionarie. Tuttavia, una lieve alterazione elettrolitica vi risparmio anche in questo caso l'aspetto medico - ci ha suggerito di trasferire il detenuto nella migliore in assoluto struttura italiana che coniugasse la sicurezza, sempre nell'ambito del 41*-bis*, con la tutela della salute. Ripetiamo sempre che, impregiudicata la certezza della pena e impregiudicata la sussistenza del 41*-bis*, la salute del la salute del detenuto, quale che sia il reato per il quale sconta la pena, è per noi un interesse primario, per ragioni etiche, giuridiche e costituzionali. Quindi, nello stesso giorno in cui è arrivata la comunicazione, peraltro non necessariamente vincolante, della struttura sanitaria di Sassari, abbiamo provveduto al trasferimento del detenuto nel carcere di Opera a Milano.

Detto questo, va aggiunto che, sempre nell'ambito del 41-*bis*, la determinazione del Governo - che che in questo momento rappresento - è in generale di mantenerlo e di non modificare minimamente la normativa che lo riguarda.

Camera, si può legittimamente discutere se sia giusto o no applicare questa norma per un certo tipo di reato piuttosto che per un altro; ma, nel momento in cui la norma esiste, la legge è uguale per tutti. Quindi non si può fare la differenza tra un 41-*bis* applicato a un terrorista anarchico rispetto a un 41-*bis* applicato a un mafioso o a un camorrista. Una volta che la legge viene applicata - e in questo caso è stata applicata su richiesta e per disposizione della magistratura ho detto prima che non esistono 41-*bis* di serie A e di serie B: la legge è uguale per tutti, quindi la disciplina che regola questo istituto - sul quale, ripeto, si può benissimo aprire una discussione quando si vuole - deve essere omogenea. Per quanto riguarda l'epilogo di questa vicenda, che si dovrebbe concludere qui per quanto riguarda la situazione su cui oggi il sottoscritto doveva riferire, cioè lo stato di Cospito, aggiungo che la situazione è stata anche aggravata, da un punto di vista generale, dall'ondata di violenze e di attentati che hanno fatto seguito a tale situazione. Stato, infatti, non può minimamente dare un segno di debolezza di fronte a qualsiasi forma di intimidazione. *(Applausi)*. La sola prospettiva, anche fallace, la sola immaginazione che lo Stato possa cedere al ricatto o alle pressioni che possono esercitarsi in varie forme per modificare le situazioni garantite e definite dalla magistratura sarebbe un'offesa non solo allo Stato di diritto, ma alla stessa sopravvivenza Questo perché, se accedessimo al principio che per un caso specifico la *pietas* prevale sul diritto, ci troveremmo un domani di fronte a tante altre situazioni analoghe che dovremmo affrontare. Se accedessimo al principio che lo stato di salute precario, anche determinato da chi lo subisce, dovesse essere una fonte di decisione di modifica del 41-*bis*, un domani ci troveremmo davanti a

Detto questo, inutile nasconderci che questo dibattito, che doveva, dovrebbe e deve essere concentrato solo sul motivo per il quale era stato chiesto e da me sollecitamente accettato - di venire il più presto possibile a riferire del caso Cospito, ha avuto una sorta di coda che si è realizzata ieri. Anche a tale proposito bisogna essere chiari. La richiesta iniziale di vari Gruppi sulla situazione di Cospito è stata in un certo senso affiancata soprattutto adesso, provenendo dalla Camera - da osservazioni che riguardano quanto è avvenuto ieri proprio alla Camera. Sono state citate informazioni che attengono a circostanze avvenute nel regime detentivo speciale di cui al 41-*bis.* È bene premettere che, in linea di principio, tutti gli atti riferibili ai detenuti in regime di 41-*bis* sono per loro natura sensibili, ragion per cui, ai fini della loro ostensione, occorre una preventiva verifica e valutazione del loro contenuto. A partire da questo dato esiste però una pluralità di aspetti che meritano doverosi approfondimenti. Questo Ministro già da ieri sera (forse avrete letto il bollettino che abbiamo emesso a tarda sera) ha disposto su questo degli accertamenti interni: bisogna comprendere di che tipo di atti si tratti; dobbiamo comprendere quale livello di segretezza abbiano, se e chi potesse averne conoscenza, se il destinatario potesse a sua volta divulgarli o condividerli con terzi. Come ho detto, nella giornata di ieri ho chiesto al mio capo di Gabinetto di ricostruire quanto è accaduto. Questi quesiti attengono a una materia che è molto complessa, delicata e suscettibile per alcuni aspetti di diverse interpretazioni. Va da sé che questo Ministro, appena esaurita questa istruttoria, è più che disponibile, anzi doverosamente si presenterà (quando sarà chiamato) nelle sedi opportune e ovviamente anche in Aggiungo, ma solo per tuziorismo, come diciamo nel gergo giuridico, che a questo si è aggiunta anche la notizia che la procura di Roma avrebbe aperto un'indagine su questo presunto reato. Noi non ci pareremo dietro la magistratura di Roma; non troveremo l'alibi dell'esistenza di questa eventuale inchiesta - se ci sarà - per dire che ce ne laviamo le mani e risponderemo soltanto all'esito di quell'inchiesta della procura; tuttavia vi sono dei limiti anche in questo caso procedurali che vanno rispettati e anche questa è una ragione per cui cerchiamo di capire quali saranno i limiti entro i quali risponderemo, quando avremo terminato quest'istruttoria, alle Camere e dove ci sarà richiesto di rispondere.

ricognizione dei fatti e soprattutto per gli elementi di chiarezza sulla vicenda che, come ha chiarito il Guardasigilli, è per sua natura molto complessa. complessa. Prima di iniziare questo breve intervento, vorrei però esprimere piena solidarietà al giornalista Stefano Fumagalli e alla *troupe* del Tg2 che ieri sera di fronte al carcere di Opera sono stati aggrediti. Io credo che la libertà di stampa non possa e non debba essere messa in discussione. Oggi in Aula affrontiamo la vicenda di Alfredo Cospito, condannato per avere gambizzato una persona nel 2012 e di avere compiuto un attentato contro la scuola dei Carabinieri di Cuneo nel 2006. Partiamo dai fatti. Cospito, che è in sciopero della fame da 105 giorni come forma di protesta contro il regime del 41-*bis,* è stato trasferito nel carcere di Opera, come il qualche minuto fa. Pur mantenendo il regime del 41-*bis,* è stato assicurato un principio che per la nostra democrazia è fondamentale: la massima tutela della salute. Su questo principio il Governo ha dimostrato coerenza e responsabilità ed è essenziale garantire le condizioni di salute del detenuto. Proprio per questo motivo, essendo venuto meno un parametro sanitario, nello stesso identico giorno in cui è arrivata la comunicazione dal carcere di Sassari, il Ministro ha disposto immediatamente il trasferimento nella struttura di Opera, dove il detenuto è monitorato con tutte le attenzioni necessarie, particolarmente dal punto di vista sanitario. Da inizio dicembre, purtroppo, stiamo assistendo invece ad atti di vandalismo perpetrati da esponenti di sedicenti gruppi anarchici che pretenderebbero l'attenuazione l'attenuazione della detenzione carceraria di Cospito. Ora voglio essere molto chiaro e su questo ritengo dovrebbe esserci una totale unità di intenti, a prescindere dallo schieramento politico, da parte di tutti noi e dal caso specifico: lo Stato non solo non deve avere nessun cedimento o fare alcuna concessione, ma non può nemmeno dare il minimo segnale di cedimento a coloro che praticano la violenza. Se lo facesse, verrebbe compromessa la credibilità del nostro sistema giudiziario, verrebbe meno lo stesso concetto, ricordato da lei prima, dello Stato di diritto: la legge è uguale per tutti. *(Applausi)*. Lo Stato di diritto si fonda per antonomasia sul principio dell'astrattezza e della generalità delle norme. Ha ragione, Ministro: apriremmo una diga che non riusciremmo più a chiudere. Lo stato di salute del detenuto va salvaguardato a prescindere e questo lo Stato lo sta già facendo. Questa linea di fermezza rispettosa della certezza del diritto non può che ricevere il nostro applauso. faccio presente che, come lei ha ricordato, i legali di Cospito hanno avviato i percorsi giuridici per impugnare o chiedere la revisione di una situazione che considerano iniqua. La decisione spetta solo, giustamente, all'autorità giudiziaria a cui la nostra stessa Costituzione garantisce completa indipendenza e autonomia e a cui noi esprimiamo massima fiducia. Cari colleghi, la politica è chiamata non ad essere spettatrice passiva, ma rispettosa del lavoro della magistratura. Non a caso, come lei ha evidenziato bene, signor Ministro, anche nel procedimento che le consentirebbe di revocare la misura del carcere duro, è comunque prevista l'acquisizione dei pareri degli organi della magistratura. È un passaggio, questo, per noi centrale. Di fronte agli attacchi ai palazzi delle diplomazie da parte di sedicenti anarchici, noi siamo convinti che da quest'Aula oggi debba levarsi un messaggio di unità da parte di tutte le forze politiche. Non possiamo abbassare la guardia nei confronti di criminalità organizzata e terrorismo, così come non possiamo minimamente strumentalizzare il dibattito politico screditando il nostro sistema giudiziario e detentivo. Questo per noi vuol dire garantismo. Per questo motivo, come Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati-UDC-MAIE, valutiamo positivamente l'intervento del ministro Nordio sulla vicenda Cospito. Signor Ministro, la sua informativa mi è parsa sinceramente non solo imbarazzante, ma anche imbarazzata. Lei non è stato in grado di informare il Parlamento, ha solo elencato una serie di fatti che conoscevamo già (bastava leggere i quotidiani in questi giorni). Avete trasformato una vicenda che si sarebbe potuta facilmente risolvere se affrontata con tempestività e se affrontata con ragionevolezza in un dramma umano e politico senza che ce ne fosse alcun bisogno. Non saremmo arrivati a questo punto se il Governo si fosse mosso per tempo. Io stesso, Ministro, avevo segnalato il problema il 3 novembre scorso, tre mesi fa, con un'interrogazione parlamentare alla quale lei non ha dato risposta per settimane; di risposte concrete, se non quella burocratica che a un certo punto è arrivata, non ne sono arrivate nemmeno in seguito, quando pure la gravità della situazione era del tutto evidente. Il Governo non ha mosso un dito; persino il trasferimento di Cospito da un carcere che non era attrezzato per prestare le cure adeguate è arrivato con immenso e inspiegabile ritardo. Soltanto un inaccettabile scarico di responsabilità, peraltro infondato, perché il Governo avrebbe potuto e dovuto intervenire e aveva gli strumenti anche normativi per farlo. Non so se questa responsabilità se questa responsabilità è una vera e propria disfatta da attribuire ad imperizia o a inettitudine, oppure a quella paura di apparire deboli, che denota però sempre massima debolezza. Quale che sia l'origine, è stato fatto un danno vero, che non coinvolge soltanto il Governo e la maggioranza, ma coinvolge lo Stato e le sue istituzioni, che rischiano, a questo punto, di apparire ciniche e inumane agli occhi di un pezzo della popolazione, oppure cedevoli e remissive agli occhi di un'altra parte del Paese. Signor Ministro, credo che ora la prima e assoluta urgenza per tutti sia impedire che questa vicenda arrivi alle estreme conseguenze e che il dramma degeneri in tragedia. Devo dirle che certamente non aiutano tutti coloro che, in questi giorni, si sono adoperati per trasformare lo sciopero della fame di Cospito addirittura in una sorta di riedizione del sequestro Moro, chiamando in causa, senza alcun fondamento, la fermezza e l'impossibilità dello Stato di trattare con chi minaccia.

non ha esitato a lanciare accuse grottesche e a diffondere informazioni riservate, di cui egli stesso non avrebbe dovuto essere in possesso. Su questo non spenderò molte parole, anche perché ho ascoltato il dibattito alla Camera dei deputati e condivido molti degli interventi che lì sono stati fatti dall'opposizione, se non che, dal mio punto di vista, è del tutto evidente che chi si comporta con questo cinismo, questa leggerezza e questa inadeguatezza non può ricoprire un ruolo delicato come la vice presidenza del Copasir *(Applausi)*. Allo stesso modo ritengo che non possa restare nemmeno per un minuto in più sottosegretario per la giustizia il deputato Delmastro Delle Vedove, che ha passato all'onorevole Donzelli le informazioni riservate perché le utilizzasse contro l'opposizione e contro quei parlamentari del Partito Democratico che hanno effettuato la visita nel carcere, nel pieno esercizio delle loro prerogative parlamentari. *(Applausi)*. Il loro è un dovere, signor Ministro, più che un diritto. Non solo li ringrazio, ma aggiungo anche che, nelle prossime ore, lo farà anche il nostro Gruppo parlamentare. Signor se immagino che lei lo sappia benissimo, che solo negli Stati autoritari si attribuiscono ai parlamentari che ispezionano un carcere le responsabilità di chi in quel carcere è detenuto. Sa dove è successo? È successo nella Turchia di Erdogan, dove hanno arrestato i deputati che andavano a vedere le condizioni di detenzione dei detenuti curdi. Succede per l'appunto negli Stati autoritari e non in quelli democratici. Lei, signor Ministro, questo lo sa meglio di me e in realtà lo ha anche ammesso nel suo intervento: spero davvero che questa consapevolezza la porti perlomeno a riconsiderare le deleghe del suo Sottosegretario. Inoltre vorrei dirle - l'ho accennato prima - che considero davvero dissennata l'evocazione di precedenti storici, che peraltro sono profondamente incisi nella memoria del nostro Paese: dissennata, controproducente e anche infondata. Credo che non sia lecito e non sia possibile alcun paragone tra la situazione di oggi e quella degli anni passati, gli anni del terrorismo, quando lo Stato - allora sì era davvero oggetto di un attacco criminale, sanguinoso e continuo. Non c'è nessuna somiglianza, nemmeno la più vaga, tra quelle organizzazioni terroristiche, quelle organizzazioni criminali e una galassia anarchica, che certamente è del tutto evidente che condanniamo, ma che è destrutturata, non piramidale e quindi evidentemente non è certo nelle condizioni di poter di poter creare gli stessi pericoli di un tempo. *(Commenti)*. In ogni caso, signor Ministro, lo Stato non deve decidere se trattare o meno, perché non c'è nessuna trattativa possibile e non c'è nessuno con cui trattare. Lo Stato deve decidere se rispondere ai valori sui quali ha giurato, se rispettare cioè le proprie leggi, oppure ignorarle, nel nome per l'appunto di una stolta inflessibilità. Il Governo deve verificare se il trattamento di Cospito in questo caso, ma di qualunque altro detenuto, sia coerente con le regole dello Stato di diritto, oppure se è una misura spropositata. L'ha spiegato stamattina Gherardo Colombo, codice e Costituzione alla mano, come la prevalenza della salute e della difesa della vita non è un'opzione, ma è ciò che la legge dispone senza limiti e senza condizioni, a maggior ragione peraltro quando appare fortemente discutibile la stessa decisione di applicare il 41-*bis* in assenza delle cosiddette possibili comunicazioni segrete tra il detenuto e l'esterno, visto che - come sappiamo tutti ormai la corrispondenza di Cospito era pubblica, con le riviste anarchiche, e bastava la censura della sua posta probabilmente, se questo era il principale dei problemi, visto che era detenuto in alta sorveglianza e non certo in libertà. Sospendere l'applicazione del 41-*bis* a Cospito non è affatto cedere a un ricatto. Mantenere quel regime, anche contro la legge, per paura di non apparire abbastanza rigidi, proprio quello invece significa cedere ad un ricatto, seppure non formalizzato. Lo Stato deve decidere sulla base di considerazioni non genericamente umanitarie, ma di rispetto sostanziale dei valori di questa Repubblica e della sua Costituzione, ma deve decidere anche - me lo lasci dire - sulla base dell'intelligenza politica, perché credo che nessuno possa onestamente ritenere che la conclusione tragica di questa vicenda, gestita davvero nella maniera peggiore possibile, agevoli la difesa dell'ordine pubblico. Sappiamo perfettamente che la realtà non è questa, di questo si tratta e di questo stiamo discutendo anche stasera; non del mantenimento o della soppressione del 41-*bis*. Naturalmente so che questo fa parte delle motivazioni dello sciopero della fame di Cospito. Io stesso ritengo anche, per aver fatto parte nella penultima legislatura, la XVII, della Commissione diritti umani di questo Senato, che sarebbe utile aprire una riflessione seria sull'articolo 41-*bis*, sulle necessità e anche sulle criticità,

non credo che si possa tacere su questo clima di lacerazione e di spaccatura che si sta cercando di creare a bella posta. Quello che dovrebbe essere un civile dibattito sul modo migliore di affrontare una specifica situazione delicata viene fatto passare per scontro tra complici della mafia o del terrorismo e difensori dello Stato. Questo è del tutto inaccettabile *(Applausi)*, non solo perché si tratta di una bugia grossolana e offensiva, ma anche e soprattutto perché da un dibattito politico ridotto a calunnia non può venire niente di buono per nessuno e soprattutto non può venire niente di buono per il nostro Paese.

ma al contempo non possiamo dirci soddisfatti di ciò che ci ha detto in merito a ciò che ne è conseguito e a ciò che si è verificato ieri nel dibattito alla Camera. Signor Ministro, lei prima ancora che uomo della politica è uomo di legge; lo dimostra la capacità con la quale ha saputo esporre tutti i fatti della vicenda giudiziaria, come ha saputo far comprendere a ciascuno di noi cosa è successo e perché Cospito è stato ristretto al regime del 41-*bis*. Per questo lei comprenderà come si renda necessario sgombrare immediatamente il campo, in questo dibattito dibattito politico, che è pubblico e che interessa chi ci ascolta, da ogni facile equivoco, cioè non spetta al Parlamento entrare nel merito delle decisioni che spettano all'autorità giudiziaria, come lei ha detto fin troppo chiaramente. Crediamo fortemente nella separazione dei poteri, primo baluardo dello Stato democratico e saldo principio della nostra Costituzione. Per questo le decisioni in merito all'applicazione del regime più severo di carcerazione non spettano a noi. E, se tali decisioni sono state assunte a seguito della riformulazione del capo di imputazione e della conseguente condanna in Cassazione, queste devono essere rispettate da noi, come Parlamento e come cittadini. Ma al tempo stesso siamo anche certi che ogni novità sarà dettata solo da una valutazione di ordine giuridico, come conviene e si attiene a uno Stato di diritto. Questa premessa era necessaria per ribadire che in alcun modo sul piatto della bilancia di questo dibattito possono finire elementi di altro tipo. E questo vale sia per lo sciopero della fame, sia per qualsiasi decisione che verrà assunta a tutela delle condizioni del detenuto. Ma questo vale, a maggior ragione, anche per le minacce e per le intimidazioni che provengono dalla galassia anarco-insurrezionalista rispetto alla decisione di confermare il regime del 41-*bis*. Le sue parole sulla conferma del 41-*bis*, sulla sua applicazione e sulla fermezza dello Stato e delle sue istituzioni in merito a tale regime ci confortano; in questo siamo assolutamente in linea con lei e con quanto ha detto prima. La vicenda Cospito non può trasformarsi ovviamente in un caso politico e guai se qualcuno, in un verso o in un altro, la intendesse in questo senso. Ma, con la stessa forza con cui crediamo nella funzione del potere giudiziario, crediamo, rivendichiamo e difendiamo le prerogative del Parlamento e dei parlamentari. Le dichiarazioni rese ieri dall'onorevole Donzelli sono molto gravi, per diverse ragioni. La prima è che nessuno, che si tratti di un parlamentare o di un semplice cittadino, può censurare un parlamentare nell'esercizio delle sue prerogative e delle sue funzioni. *(Applausi)*. In questo, signor Ministro, la visita nelle carceri, la visita ai detenuti per l'accertamento delle loro condizioni di vita e di salute non sono soltanto una funzione, ma sono prima di tutto un dovere di ogni parlamentare. L'onorevole Donzelli non ha mancato di rispetto di rispetto solo alle opposizioni; ha mancato di rispetto all'intero Parlamento. *(Applausi)*. Questa offesa è stata aggravata Questa offesa è stata aggravata dal volgare e irricevibile accostamento tra i parlamentari andati in visita in carcere al fenomeno della mafia e del terrorismo. *(Applausi)*. Tanto già basterebbe Tanto già basterebbe a censurare le sue parole, se non fosse che al peggio purtroppo non c'è fine. L'onorevole Donzelli, Vice Presidente del Copasir, ha alimentato un inaccettabile accostamento. E lo dico

e la lotta, ad opera di elementi anarchici e personaggi mafiosi, al regime carcerario del 41-*bis*. Per fare questo accostamento, per creare questa confusione questa suggestione in chi ha ascoltato il suo intervento, si è avvalso di un rapporto che riferiva in merito ad alcune intercettazioni ambientali tra Cospito e detenuti condannati per mafia e ristretti anch'essi al regime del 41-*bis*. Le ammissioni successive del sottosegretario Delmastro Delle Vedove, che poi si scopre essere pure coinquilino dell'onorevole Donzelli, sul fatto che sia stato lui stesso a rivelargliele getta una pesante ombra sull'adeguatezza di entrambi a ricoprire i delicati incarichi di Sottosegretario e di di Sottosegretario e di Vice Presidente del Copasir. *(Applausi)*. Le conseguenze di questa latitanza del senso delle istituzioni e del rispettivo ruolo istituzionale sono semplicemente catastrofiche. Signor Ministro, io me lo chiedo e glielo chiedo: c'è consapevolezza che in questo modo si è probabilmente bruciato un filone investigativo? *(Applausi)* Che si è messo a repentaglio il lavoro di intercettazione di intercettazione preventiva delle conversazioni di detenuti ad alto indice di sorveglianza, che viene condotta generalmente dagli agenti del gruppo operativo mobile della Polizia penitenziaria? Con quale spirito un qualsiasi funzionario dei nostri Servizi condividerà le informazioni coperte dal segreto nelle audizioni al Copasir, se poi sa o è venuto a conoscenza o con rammarico ha dovuto apprendere che il Vice Presidente del Copasir è stato pronto a farne materia di chiacchera e arma di intimidazione politica agli avversari? Signor Ministro, noi ci auguriamo che le iniziative da lei annunciate sull'accertamento dei fatti portino a un riscontro concreto, in tempi rapidi. Ma pensiamo che in un Paese serio le dimissioni di persone che hanno dimostrato di non saper maneggiare informazioni sensibili sarebbero già sul tavolo. *(Applausi)*. Qui infatti il tema vero non è l'ubriacatura da potere, come ha scritto qualcuno, o uno sgangherato tentativo di distrarre l'attenzione dai magri risultati dei primi cento giorni di governo. Una vicenda di enorme delicatezza, che avrebbe dovuto richiamare le istituzioni e i suoi rappresentanti ad un profilo austero, anche sulla comunicazione delle decisioni assunte, è stata maneggiata con grande spregio delle istituzioni parlamentari e deplorevole incuria del lavoro svolto dalle Forze dell'ordine e da tutti coloro che operano per garantire la sicurezza dello Stato. In conclusione, signor Ministro, ci sia consentito aggiungere che anche questa vicenda dimostra ancora una volta lo stato di dissociazione esistente tra chi governa e se ne sta chiuso nei palazzi dorati e i cittadini italiani, stretti nella morsa di una crisi economica sempre più forte, con un Meridione che diviene sempre di più attacco di scelte politiche improntate alla disuguaglianza e alla cinica sottrazione di risorse. I cittadini attendono risposte alle domande fondamentali della nostra vita quotidiana: sul lavoro, sull'occupazione, sulla retribuzione, sulla pensione, sulla scuola, sulla giustizia, sulla sanità, sulla salute. Invece, si trovano costretti a assistere a scomposte dichiarazioni del Vice Presidente del Copasir che divulga informazioni riservate per attaccare gli avversari politici. Anche per questo, signor Ministro, non ce ne voglia, ma una parola da parte della Presidente del Consiglio sarebbe stata gradita. *(Applausi)*. A meno che la Presidente

noi abbiamo apprezzato il tono civile ed istituzionale che il signor Ministro ha portato in quest'Aula, le parole che ha detto e potrei dire, con un sorriso, anche le parole che non ha detto, che non ha voluto dire, che non ha potuto dire. Effettivamente, questa vicenda è surreale. Non è la prima vicenda surreale di questo inizio di legislatura. Sembriamo specializzati nell'inseguire gli argomenti che i media o i *social* ci indicano. Siamo partiti con il *rave party*; poi ci siamo dedicati per un mesetto al Pos, peraltro senza alcun atto formale su questo; ci siamo buttati per una decina di giorni sui cinghiali e poi siamo tornati sul MES. Avevamo l'occasione finalmente di festeggiare un grande risultato: la cattura di Matteo Messina Denaro, che è un grande risultato dello Stato, delle istituzioni, di tutti noi insieme. *(Applausi)*. Questo clima, però, ieri è stato rotto, proprio sul voto unanime sulla Commissione antimafia, da un intervento sguaiato e del tutto fuori luogo dell'onorevole Donzelli. Tuttavia, questo pone un tema politico, che affronterò nel finale. Prima faccio tre brevissime considerazioni. La prima: il ministro Nordio oggi è stato bravo nel ribadire e spiegare che il cardine della democrazia liberale è il principio della separazione dei poteri. Io sono tra quelli che in questa Aula è venuto a dire che i magistrati non potevano invadere il terreno della politica laddove si permettevano di decidere le forme organizzative della medesima. Allo stesso modo, sento il dovere di dire che sul destino di un detenuto, che è passato da tutti i gradi di giudizio, non in tutti i processi, ma che è comunque affidato alla giustizia italiana, il Parlamento non ha un compito di decisione come se noi potessimo intervenire sul singolo caso perché presi dal richiamo mediatico per cui ciascuno, in questo gigantesco bar dello sport che è diventato la politica, deve dire tutto su tutto. Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu, spiegava che il cardine della democrazia liberale è proprio la separazione dei poteri. Allora, i parlamentari facciano i parlamentari, facciano le leggi e rispettino i magistrati, alcuni dei quali sono anche oggetto di minacce, come ella, signor Ministro ha ricordato; magistrati che hanno il compito e il dovere di assicurare alla giustizia i singoli. Secondo punto: ma allora noi che ci stiamo a fare? Noi possiamo mettere in discussione le leggi e possiamo cambiarle. Questo è legittimo per un Parlamento. Io non mi straccio le vesti se qualcuno viene qui e chiede di cambiare delle leggi esistenti. Penso, però, che non si possa fare quando qualcuno ci costringe a discuterne facendo saltare le auto dei nostri diplomatici all'estero; quando qualcuno ci costringe a farlo aggredendo magistrati, aggredendo le Forze dell'ordine. Non si fa così una discussione. *(Applausi)*. Una discussione civile sul 41-*bis* si può fare. Io credo che il 41-*bis* abbia salvato il Paese. Ho una mia opinione, che magari non è condivisa da tutti. Credo che la legislazione speciale italiana - ancora prima sul terrorismo e poi sulla mafia - abbia permesso a questo Paese di vincere vere e proprie emergenze.

è stata la politica a sconfiggere la mafia; non è vero, come ci hanno raccontato per trent'anni, che la politica era schiava della mafia. Certo, ci saranno state responsabilità di singoli, ma è la politica, con il ministro Martinazzoli, che costruisce l'aula bunker per Giovanni Falcone quando questi gli chiede di fare il più grande processo della storia penale del paese, che ha vinto in quel passaggio. E quando taluni magistrati - e correnti giudiziarie attaccano il giudice Falcone, è il ministro della Repubblica Martelli che lo chiama a Roma dandogli la possibilità di essere in prima linea nel combattere la mafia. *(Applausi)*. E quando Falcone viene ucciso dalla mafia, è in quel momento lì che nasce il 41-*bis* per tentare di distruggere la mafia; cosa che sta avvenendo, alla faccia di tutti quelli che ci raccontano che ci sono state trattative più o meno fantasiose, che vengono smentite dalla Cassazione e che permettono a qualche ex magistrato di fare carriera e di entrare in questo Parlamento, ma che non corrispondono alla realtà dei fatti. *(Applausi)*. È stata la politica con i propri rappresentanti a fare la legislazione speciale, e questo va spiegato a chi ancora continua a non capirlo. Volete cambiare il 41-*bis*? Ditelo. Io sono contrario. *(Applausi)*. Sono contrario in questo momento, ma rispetterò l'opinione di chi vuole cambiarlo. Il 41-*bis* è stata la grande vittoria della politica contro la criminalità organizzata. Su questo c'è il terzo punto, che riguarda voi, colleghi della maggioranza.

le sue - perché quando vai a votare la legge istitutiva della Commissione antimafia non ti metti ad attaccare gli avversari accusandoli di non essere lo Stato. *(Applausi)*. Sapete chi non è lo Stato? Non è lo Stato chi in questo Paese utilizza materiale riservato per attaccare gli avversari:

di casa che si condivide, ma c'è un rispetto delle istituzioni che, prima o poi, vi porterà a chiedere il conto di quello che avete fatto in questo passaggio. Vengo al punto fondamentale, ed è un punto politico. Ha ragione

Noi siamo dalla parte della legalità, siamo dalla parte della giustizia. Vi diciamo, allora: c'è o non c'è un contrasto tra l'idea liberale di una destra che sulla giustizia ha una visione garantista - garantismo non vuol dire buonismo, attenzione, non vuol dire abolire il 41-*bis* abolire il 41-*bis* - e chi invece ha un'idea giustizialista cresciuta nella visione forcaiola che ieri è stata espressa? Fino ad oggi la presidente Meloni, molto abile - lo sottolineo - è stata brava nel far capire che eventuali difficoltà interne alla propria maggioranza derivassero dai propri alleati, e su questo ha avuto buon gioco, talvolta a lamentarsi della Lega, talvolta di Forza Italia: è legittimo, è il gioco delle parti, l'abbiamo fatto tutti; è politica. Stavolta il problema è un altro: tra il Ministro della giustizia, un galantuomo liberale eletto con Fratelli d'Italia, e due colonne di Fratelli d'Italia che dicono esattamente il contrario di quello che il Ministro ha detto fino ad oggi. *(Applausi)*. C'è allora un punto politico che vorrei che il Parlamento affrontasse, anziché continuare a inseguire costantemente le discussioni del *day by day:* via la discussione sul singolo detenuto; tocca ai magistrati decidere. Volete intervenire sul 41-*bis* e parlarne? Noi ci siamo; siamo perché lo Stato vinca e lo faccia attraverso anche la legislazione speciale. Nelle università americane studiano la nostra legislazione speciale su terrorismo e mafia; altro che fandonie sulle trattative di qualche ex pm in cerca di ruolo politico! Alla luce di questo, però, voi della maggioranza abbiate il coraggio di dire che questo tema prima o poi dovrete scioglierlo: o si sta dalla parte del garantismo, del principio della democrazia liberale, di ciò che il ministro Nordio ha spiegato, o si continua a fare quello che nei primi cento giorni quello stesso Sottosegretario - che ha passato gli atti in modo a dir poco maldestro - ha fatto, facendo costantemente il controcanto. Signor Presidente, ho concluso. È un tema politico, finalmente, vivaddio. C'è una grande questione che riguarda questa maggioranza così solida nei numeri: volete avere una visione dello Stato moderno, con una giustizia liberale capace di dimostrarvi una forma di partito conservatore moderno, o pensate di rincorrere il giustizialismo forcaiolo di Donzelli e del Sottosegretario? A voi la scelta. Noi stiamo dalla parte del Ministro, della Costituzione, della giustizia.

Ministro Nordio, prendiamo atto della sua relazione e la ringraziamo per essere qui in Senato a renderla a questo consesso; l'abbiamo giudicata puntuale sotto il profilo giuridico-politico e anche rimarchevole per la solerzia con cui lei si è attivato ed è venuto in Senato.

dal ministro Nordio e che è stato destinatario di minacce di morte, ma anche a tutti quei magistrati e soggetti dello Stato che pure sono stati destinatari di minacce in questi anni da parte della galassia anarchica, nonché alla *troupe* del TG2 e del giornalista Fumagalli, che ieri è stato oggetto di un'aggressione nei pressi del carcere di Opera. Partiamo

va premesso che maggiore prudenza nelle esternazioni in questioni così delicate come il 41-*bis* sarebbe stata più opportuna. *(Applausi)*. da giuristi comprendiamo perfettamente la necessità di verificare la natura delle informazioni che sono state diffuse ieri sera alla Camera dall'onorevole Donzelli, perché è del tutto evidente che va preliminarmente chiarito se si trattava di dati segreti, dati riservati o dati liberi: questo è preliminare a qualsiasi valutazione. Le conseguenze giuridiche e politiche sarebbero evidentemente diverse in relazione alla diversa natura dei dati resi noti e dalle diverse modalità di acquisizione. Tale accertamento spetta *in primis* a lei e agli uffici del Ministero. La conosciamo come un galantuomo e un Ministro e magistrato integerrimo. In questo primo scorcio di legislatura abbiamo più volte espresso totale fiducia nel suo operato e la riconfermiamo stasera. Diciamo subito che accetteremo con serenità tutte le decisioni che lei andrà ad assumere e i giudizi che andrà ad esprimere. Veniamo al caso Cospito, così dedicato sotto i profili giuridici, etici e anche morali. Forza Italia innanzitutto ribadisce che il 41-*bis* non deve essere oggetto di una trattativa con chi pratica la violenza. Abbiamo parlato tante volte - il più delle volte a proposito della trattativa Stato-mafia. Ebbene, pensare che oggi possiamo modificare il 41-*bis* a causa degli attentati o delle intimidazioni della galassia antagonista o dello sciopero della fame di Cospito sarebbe inaccettabile, costituirebbe un errore e anche, come giustamente diceva il Ministro, un precedente gravissimo e inaccettabile. Il 41-*bis* ha funzionato e continua a funzionare, per interrompere e recidere in modo netto i legami tra i vertici delle organizzazioni criminali e i loro sodali. Va detto e va ricordato - e lo diciamo con orgoglio - che il 41-*bis* è stato messo a regime e reso permanente proprio dal Governo Berlusconi nel 2002, e poi è stato rafforzato anche nel 2009. Di questo, noi di Forza Italia siamo particolarmente orgogliosi. Modificarlo oggi, sotto il ricatto dello sciopero della fame di Cospito o delle violenze degli anarchici, è un'ipotesi che rigettiamo senza alcuna esitazione. Lo Stato deve essere fermo e dare l'impressione di non essere diviso al proprio interno, pena la sua permeabilità e la sua debolezza. signor Ministro, su questo punto perfettamente d'accordo con lei: il 41-*bis* non si tocca. Ciò detto, vanno precisati alcuni aspetti. Il primo l'applicazione o meno del 41-*bis* è un atto giurisdizionale, un atto tecnico non politico. Allora, colleghi del Partito Democratico, consentitemi di stupirmi dell'intervista che oggi ha rilasciato l'onorevole Orlando sul quotidiano «Domani», in cui in buona sostanza accusa l'ex ministra Cartabia di aver esagerato applicando il 41-*bis* a Cospito quando: «si poteva pensare ad un regime intermedio». quale doveva essere il regime intermedio. All'epoca la Ministra, per quanto risulta agli atti (credo che nessuno li abbia smentiti), ha firmato su richiesta concorde, come ci ha detto anche il ministro Nordio, della direzione distrettuale antimafia di Torino e della Direzione nazionale antimafia, che dimostrarono in modo chiarissimo e equivocabile che Cospito aveva fatto pervenire dal carcere «documenti di esortazione alla prosecuzione della lotta armata di matrice anarco-insurrezionalista». Non ci sono pertanto dubbi sulla correttezza ministeriale. Da ex Ministro della giustizia l'onorevole Orlando dovrebbe sapere che il Ministro, quando firma o revoca il 41-*bis,* lo fa sulla base delle risultanze della magistratura; il suo è un atto tecnico, vincolato, non discrezionale,

del tutto evidente che Cospito, come testimonia l'intervista della sorella apparsa oggi sul quotidiano «La Repubblica», va cercando la bella morte, che lo consegnerebbe alla storia e lo trasformerebbe in un simbolo. Questa eventualità a nostro giudizio va sventata con ogni mezzo. Oggi Cospito non è un individuo libero, ma liberamente ha scelto la sua sorte: il suo corpo e la sua salute sono affidati allo Stato e lo Stato dovrà fare di tutto - lo ripeto: di tutto - per evitare che egli muoia in carcere, financo Non possiamo permetterci che lui diventi il Bobby Sands italiano, legittimando una nuova figura patologica di eroismo. In terzo luogo,

se queste dichiarazioni, invece di renderle Gherardo Colombo, le avesse rese il presidente Berlusconi, cosa sarebbe successo? Quali ululati si sarebbero alzati dai banchi del MoVimento 5 Stelle? Quanta indignazione sarebbe stata manifestata - credo - anche all'interno del Partito Democratico? Noi sappiamo bene che essere garantisti non è facile: noi lo siamo sempre stati a 360 gradi, non andando da una parte o dall'altra a seconda delle convenienze politiche del momento. Nell'intervista che oggi ha rilasciato l'ex ministro Orlando si coglie un senso di critica al 41-*bis.* Allora io chiedo ai rappresentanti condividono quelle posizioni, se pensano che il 41-*bis* vada modificato. Tuttavia una premessa deve essere chiara: l'ha detta bene il Ministro e io la sposo totalmente. La legge è uguale per tutti. Non possiamo pensare di modificare il 41-*bis* magari per gli anarco-insurrezionalisti e lasciarla invece per i mafiosi

perché è troppo facile fare i garantisti a tempo alterno. Forza Italia è riuscita - credo lo abbia dimostrato in ormai trent'anni di attività parlamentare - a mantenere sempre la barra dritta

apre una nuova finestra") *(M5S)*. Ci vuole una bella faccia tosta come quella del senatore Renzi per qualificare il 41-*bis* come una vittoria della politica.

Senatore Scarpinato, non si è avvertito da qui nessun disturbo e la prego di rivolgersi alla Presidenza e, attraverso la Presidenza, se vuole, agli altri colleghi, magari usando, se ritiene, un linguaggio consono. SCARPINATO *(M5S)*. Spero che potrò recuperare questi secondi. Il senatore Renzi ignora che la legge che introdusse il 41-*bis* è una legge sporca di sangue, perché è una legge che fu introdotta esclusivamente con il sangue versato da Paolo Borsellino e dai cinque agenti della scorta, trucidati nella strage di via D'Amelio, e con l'indignazione popolare che ne seguì, che costrinse un Parlamento riottoso, che non voleva approvare il 41-*bis* definendo forcaioli e giustizialisti coloro che lo proponevano, ad approvarlo. Non fu, quindi, una vittoria

È una legge sporca di sangue e non si può definire una vittoria della politica. Vengo qui al caso Cospito. Noi siamo veramente preoccupati, signor Ministro, per l'acuirsi della grave sindrome dello sdoppiamento della personalità da cui lei è chiaramente affetto e di cui abbiamo già colto in passato sintomi evidenti. Avevamo già capito che lei al mattino è un feroce giustizialista, quando si tratta di introdurre con decreto-legge reati come quello di *rave*, per i quali aveva previsto intercettazioni, misure di prevenzione antimafia e pene severissime, e al pomeriggio si trasforma in un garantista, quando si tratta di reati di colletti bianchi, proponendo di abolire intercettazioni e reati come abuso d'ufficio e traffico di influenza. *(Applausi)*. Oggi abbiamo scoperto che lei al mattino è un Ministro estremamente bellicoso e rigoroso, quando si tratta di sanzionare indebite fughe di notizie di intercettazione giudiziaria, definite da lei porcherie per le quali ha più volte dichiarato che sarebbe stato inflessibile, avrebbe usato il pugno di ferro, avrebbe attivato i suoi poteri ispettivi per accertare le responsabilità, anche se - come lei ha acconsentito - erano in corso indagini per reato di agevolazione di segreti d'ufficio, perché il Ministro può fare ispezioni. Poi - sintomo evidente di sdoppiamento della personalità - si trasforma nel tardo pomeriggio in un Ministro che si mette la coda tra le gambe e si arrampica sugli specchi farfugliando scuse improbabili, quando si verificano gravissime fughe di notizie - porcherie, per usare le sue parole - che provengono direttamente dagli uffici del DAP e in particolare dal sottosegretario per la giustizia con delega al DAP Delmastro Delle Vedove. La informo, signor Ministro, che il suo Sottosegretario ha bellamente confessato alla stampa di aver rivelato a un suo compagno di partito, coinquilino, onorevole Donzelli, notizie acquisite grazie al suo ruolo istituzionale e di cui non aveva alcuna disponibilità personale, di estrema rilevanza penale e che dovevano restare segrete e cioè che agenti della Polizia penitenziaria avevano accertato che vertici mafiosi stavano cavalcando e strumentalizzando la protesta di Cospito per ottenere l'abolizione del 41-*bis.* Notizie che lei, come ex magistrato, sa benissimo che dovevano essere coperte dal massimo segreto e trasmesse immediatamente alla procura nazionale antimafia, che le avrebbe trasmesse alla procura della Repubblica, per attivare indagini urgenti e segretissime, con intercettazioni ambientali all'interno del carcere. Un Sottosegretario con delega al DAP che non è in grado di capire la segretezza delle notizie che ha acquisito e di mantenere la segretezza di queste notizie non è in grado di continuare a svolgere il suo ruolo. Come se non bastasse, l'onorevole Donzelli ci ha fatto assistere, ieri, alla Camera dei deputati, alla consumazione di un reato in flagranza: la rivelazione di segreti di ufficio. Ha cioè rivelato alla Nazione, notizie che aveva indebitamente acquisito e che dovevano restare segrete, compromettendo così definitivamente l'esito di indagini giudiziarie importantissime. ciò, per di più, solo per sferrare un attacco politico a componenti dell'opposizione: altro evidente segno di inadeguatezza

come è accaduto, ma non ha neppure la forza politica e l'autorevolezza personale per fare l'unica cosa che avrebbe dovuto fare, ovvero chiamare l'onorevole Delmastro Delle Vedove e invitarlo gentilmente a rassegnare le dimissioni, per tutelare il decoro delle istituzioni. Oggi invece viene qui a prendere tempo, a nascondersi dietro il corso delle indagini e a dare motivazioni implausibili. Abbiamo quindi un grave problema, signor Ministro: lei non è in grado di assolvere le sue funzioni e, nell'interesse dello Stato, dovrebbe valutare se rassegnare le dimissioni. vi prego di non adeguarvi ad un andazzo che non mi piace: quello dell'ululato. È

il fatto che, prima di prendere una decisione, il Ministero, a norma di legge, deve attendere i pareri che devono arrivare dalla procura generale della corte d'appello di Torino e anche dalla Direzione nazionale antimafia, seguendo quindi una procedura. Questa è una risposta chiara e corretta, rispetto ad una richiesta di revoca che è arrivata al Ministero. Quindi, ha spiegato bene la procedura e ha chiarito in modo evidente che il trasferimento al carcere di Opera, uno dei migliori d'Italia - ci tengo a sottolinearlo - è una garanzia ulteriore per il detenuto. Ha dunque messo in evidenza alcuni principi,

perché è giusto essere garantisti, ma bisogna anche fare in modo che lo Stato mostri la sua fermezza: di questo siamo assolutamente contenti e soddisfatti. *(Applausi)*. Su quello che è accaduto ieri alla Camera ha sostanzialmente detto che c'è un approfondimento in corso e quindi attendiamo l'approfondimento e, anzi, il fatto stesso che il Ministero non voglia lavarsene le mani, come qualcuno magari poteva immaginare, è invece un segno di forte responsabilità. La maggioranza deve anche trarre esperienza da queste situazioni che si vengono a creare, cercando il più possibile di evitare quelle che sono delle provocazioni; soprattutto sul tema della giustizia, cerchiamo tutti di abbassare i toni e di affrontarlo con un con un approccio più tranquillo e moderato, ma mi rivolgo a tutti, perché in queste settimane sono state tante le occasioni per alzare i toni su tale questione. Evitiamo di porre la solita questione dello scontro tra politica e magistratura; basta con questi vecchi *cliché*, perché altrimenti davanti all'opinione pubblica non saremo mai più in grado di essere credibili e la gente andrà sempre meno a votare. Quindi, l'invito davvero rivolto a tutti è a una maggiore responsabilità e al confronto.

sostanzialmente di far intendere che si sta dalla parte di anarchici che stanno manifestando, anche con alcuni episodi di violenza, contro il 41-*bis*. *(Applausi)*. Un atto di responsabilità da parte di tutti, abbassando i toni, è la strada giusta per un confronto e una dialettica che possano anche portare nel tempo ad una serie di riforme, ovviamente su tantissimi campi, perché sono tanti i campi sui quali dovremo discutere. Però cambiamo un po' l'atteggiamento, perché andando avanti così sarà molto difficile da parte di tutti essere credibili - ripeto - agli occhi dell'opinione pubblica.

ministro Nordio, stando all'intervento che ha fatto noi saremmo la coda, perché in realtà noi abbiamo chiesto il suo intervento anche in questo ramo del Parlamento per porre l'attenzione su quello che è successo ieri alla Camera, che per noi - glielo dico con grande convinzione - è una questione che riguarda tutto il Parlamento, il rispetto delle istituzioni e la stessa qualità della nostra democrazia. Non so come dirglielo, Ministro: sono state mosse accuse gravissime ieri, rivolte a deputati e a un senatore del Partito Democratico, il senatore Verini, a cui va tutta la nostra solidarietà e il nostro abbraccio. Rispetto a queste accuse, per cui è stato convocato per competenza anche il gran giurì della Camera, appunto il luogo dove sono state mosse, ogni parlamentare deciderà poi come agire. Però, Ministro, io volevo attenermi ai fatti, quelli che lei si è dimenticato di raccontarci oggi in questa sede e nella sua relazione; li ha completamente ignorati, perché guardando solo ai fatti quello che emerge è una vicenda gravissima. Il fatto che un parlamentare della Repubblica, coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, uomo di fiducia della Presidente del Consiglio, l'onorevole Donzelli, venga in Aula ad accusare il Partito Democratico, ventilando contiguità e ambiguità su terrorismo e mafia, è di una gravità inaudita. Sono accuse pesanti, rivolte per il solo fatto che parlamentari autorevoli e seri della Commissione giustizia, hanno esercitato il loro diritto, ma anche direi il loro dovere, di andare in carcere ad accertarsi delle condizioni di salute di un detenuto, agendo nell'ambito delle loro prerogative parlamentari, che lei - lo ammetto - ha riconosciuto, Ministro, sconfessando pubblicamente Donzelli da questo punto di vista, ma che evidentemente certa destra non conosce o preferisce ignorare. *(Applausi)*. Nessuno di noi - lo dico per chiarezza, così sgombriamo il campo da tutti gli equivoci di questa discussione ha mai messo in dubbio l'articolo 41-*bis*. E mi fermerei qui, rispetto a questo tema. Siamo andati in carcere a verificare le condizioni di salute di un detenuto, chiedendo che fosse trasferito in un luogo più idoneo a sua tutela, tutela, per la sua salute, cosa che il Governo ha fatto, purtroppo non puntualmente, perché ha atteso tanto tempo. Forse, se il Governo avesse agito prima, anche un certo clamore si sarebbe attenuato; noi era da tempo che lo dicevamo. La cosa però ancora più grave e intollerabile è che le rivoltanti accuse verso il Partito Democratico siano state fatte utilizzando informazioni riservate, che non erano accessibili ad alcun parlamentare, a differenza di quello che ha detto più volte l'onorevole Donzelli; informazioni fornite dal sottosegretario per la giustizia

questo stesso Sottosegretario, cioè che in fondo quelle informazioni riservate e non divulgabili sono state trasmesse solo oralmente; gliele ha raccontate. Poi si vede che il caro Donzelli ha una memoria di ferro, perché invece ieri le ha lette dettagliatamente; ha letto proprio quelle che potevano essere addirittura delle trascrizioni. Ciò significa che quei documenti li aveva visti, li avrà memorizzati, avrà studiato benissimo. Fatto sta che quei documenti lui li ha visti; e sono documenti che sono nel suo Ministero, Ministro, sono al Ministero della giustizia. il suo Sottosegretario ha detto oggi che è disponibile a dare tutte le informazioni di questo tipo a chiunque le chieda. Lei, Ministro, cosa ne pensa? Almeno questo qui ce lo poteva dire, perché ci sono delle agenzie di stampa; almeno questo ce lo poteva dire. Vorrei chiederle anche se le sta bene che il suo Sottosegretario, sempre nelle agenzie (quindi lo ha detto lui), abbia dichiarato legittimo trasmettere informazioni riservate non solo ai deputati, ma anche agli amici. agli amici. Io mi chiedo cosa pensino i colleghi della maggioranza dell'onorevole Donzelli. Agli amici. Delle Vedove nel suo racconto - perché oltretutto sono stati incredibilmente loquaci in queste due giornate - ha dichiarato che non sapeva che l'onorevole Donzelli avrebbe fatto un intervento utilizzando quelle informazioni. Allora è del tutto evidente che si trattava di informazioni che non andavano divulgate. E almeno qui non l'ha fatto lei, Ministro, ma il sottosegretario Delmastro Delle Vedove ci ha fatto capire qualcosa di questa vicenda. Ma è questa la serietà con cui si può affrontare un incarico istituzionale? Ministro, lei si sente sicuro con questo Sottosegretario? Si sente sicuro di potergli affidare incarichi? Si sente sicuro che quel vincolo di riservatezza possa essere garantito? E noi, colleghi, possiamo sentirci sicuri con un Vice Presidente del Copasir che utilizza informazioni riservate non solo con superficialità, ma per colpire le opposizioni? *(Applausi)*. Pensiamo che sia una cosa legittima? Lo dico ai colleghi del Parlamento. Qui non c'entra il colore politico, non c'entra l'appartenenza; c'entra il nostro ruolo, Ministro, ricapitolando, c'è un Sottosegretario che fornisce informazioni riservate a un suo compagno di partito, che è anche coordinatore nazionale del primo partito di maggioranza, che è uomo di fiducia della *Premier*, che utilizza queste informazioni riservate per colpire indegnamente l'opposizione.

che quello che è accaduto ha messo in discussione lo Stato di diritto, le regole su cui si basano le istituzioni democratiche. che quanto accaduto mette una mina pesante su quel rapporto di fiducia che comunque ci deve essere nelle relazioni tra maggioranza e opposizione, perché è su quelle relazioni e su quella forza

perché noi già oggi pretendiamo una parola chiara e una risposta politica dal Presidente del Consiglio. Qual è la cultura istituzionale che il Presidente del Consiglio chiede ai membri del suo Governo? È quella dell'immagine che abbiamo visto ieri e oggi con il sottosegretario Delmastro Delle Vedove? È questa la cultura che vuole il Governo e che ha in mente Giorgia Meloni?

e della volontà di far uso politico e strumentale di informazioni riservate, è stato messo a rischio il lavoro quotidiano che le istituzioni fanno

l'informativa del ministro Nordio si è svolta su tre piani: il primo è sulle ragioni e il fondamento dell'applicazione del regime di carcere duro di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario al terrorista condannato per associazione a delinquere con finalità di terrorismo, signor Cospito. Su questo punto, senatrice Malpezzi, nessun balbettio, nessun silenzio imbarazzato. Su questo punto, parole chiare: il 41-*bis* è uno strumento fondamentale nella lotta alla mafia e al terrorismo e nessun sciopero della fame può metterlo in discussione, con buona pace, con buona pace, cari colleghi della sinistra, di quella sinistra mediatica e politica che, invece, il 41-*bis* lo mette in discussione. Eccome! Gherardo Colombo, Massimo Cacciari, Roberto Saviano, l'onorevole Orlando l'onorevole Provenzano, a vario titolo e con vari argomenti hanno tutti messo in discussione *(Applausi)*. Noi stiamo col Ministro. Noi stiamo con le vittime dei reati. Noi stiamo con la gente perbene. Noi stiamo con la legalità. Fatevene una ragione. Chi parla di dramma umano, senatore De Cristofaro, chiedendo la sospensione, se non la revoca del 41-*bis*, non tiene conto di un fatto. Cospito non sta digiunando per se stesso; non sta protestando per se stesso. Lo ha dichiarato apertamente: anche se fosse revocato il 41-*bis* nei suoi confronti, continuerebbe la sua battaglia. Si considera un prigioniero politico. E quando il senatore De Cristofaro dice che non c'è alcun collegamento fra la posizione di Cospito e quella delle brigate rosse, lo dovrebbe spiegare a Cospito. Cospito. Cari colleghi, leggo: «Contributo per l'assemblea del 9 giugno 2019 a Bologna», da un sito anarchico, firmato Alfredo Cospito, sempre per l'anarchia,

i compagni delle BR, compagni comunisti ed un nostro compagno Marco che si trova ad Alessandria». Prendete atto di queste parole di vi prego. Prima ho sentito parole pesanti, forti - senza che nessuno abbia disturbato - legittimamente espresse dai vari oratori.

quando ha detto che qualche ex magistrato vagheggia trattative e terzi livelli inesistenti e su questi teoremi, smentiti da tutte le sentenze,

uno di costoro è seduto due file sotto di lei.

cari colleghi - Donzelli ha detto quello che è evidente a qualsiasi persona di buonsenso *(Applausi)*. Qualcuno ha dubbi che la mafia avrebbe strumentalizzato e si sarebbe infilata in questa breccia che anche voi avete contribuito, magari involontariamente, ad aprire?

Nessuno può censurare un intervento sgradito,

credevo che in quest'Aula ci fosse libertà di opinione.

l'onorevole Donzelli ha parlato alla Camera facendo quelle straordinarie rivelazioni, cioè scoprendo l'acqua calda, su «la Repubblica»,

quello che ha detto l'onorevole Donzelli è vero o non è vero? *(Applausi)*. È questo che interessa alla gente. C'è una rivelazione del segreto d'ufficio? Ci sono le indagini interne in corso. Avete fatto anche un esposto alla magistratura, che farà i suoi accertamenti. Complimenti al vostro garantismo *(Applausi)*, perché il vostro garantismo vi ha trasformato in accusatori e in giudici e avete già emesso la sentenza. Altro che balbettio del ministro Nordio. Il ministro Nordio ha detto: appena avrò delle certezze, perché il tema è delicato e complesso, verrò in Parlamento a riferirle. Questo è un vero Ministro. terzo livello del suo intervento, ministro Nordio, il Partito Democratico si è sentito offeso dalla domanda del collega Donzelli. una domanda retorica che in realtà non voleva dire - come qualcuno lo ha accusato - che il PD sta con la mafia. Non era questo ovviamente il senso dell'intervento dell'onorevole Donzelli. Fate almeno credito alla sua intelligenza. Voleva dire esattamente quello che ho detto prima: ma non vi rendete conto, colleghi, che andando in carcere il 12 gennaio a trovare Cospito avete aperto una voragine? E l'avete aperta alla mafia. *(Applausi)*. Io sono d'accordo che si possa andare in carcere, ci mancherebbe altro. In questo Parlamento pensavo che ci fosse la libertà di opinione. Evidentemente, per la sinistra la libertà di opinione ce l'ha solo il senatore Scarpinato quando ci insulta. Volete andare in carcere a verificare le condizioni di salute di un detenuto? È encomiabile, ma vi faccio una domanda: una una volta che avete verificato questo, perché dovete tenere una conferenza stampa di fronte al carcere criticando, con le parole di Orlando, il 41-*bis*? *(Applausi)*.

con una modesta osservazione: io ho ascoltato in quest'Aula con rispetto, pur non condividendole, frasi molto più gravi di quelle che ieri il deputato Donzelli ha

che nella maggioranza del *premier* Meloni c'è un partito il cui *Premier* ha avuto a lungo rapporti e contatti con la mafia.

questo - avete applaudito Scarpinato quando diceva queste cose! Andate a rivedervi i filmati! Non tutti, ma una parte dei colleghi del PD lo hanno intrattenuto. Vi sentite offesi, ma pensate a quanti insulti ci avete rivolto in tutti questi anni. Ci sarà un giurì d'onore che giudicherà

perché si è sentito chiamato in causa dal mio passaggio sui magistrati che, in nome di una fantomatica trattativa smentita dalla sentenza di Corte di cassazione, hanno costruito una carriera in magistratura e poi in politica. Vorrei che restasse agli atti del verbale che effettivamente mi riferivo esattamente a Roberto Scarpinato *(Applausi),* al quale vorrei ricordare che, prima di venire a dare della faccia tosta ai colleghi, dovrebbe spiegare non solo le sue strane frequentazioni con il dottor Palamara, ma anche il suo atteggiamento del tutto folle nei confronti delle istituzioni di questo Paese, come sa il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano.

possano esprimersi senza essere disturbati, qualunque sia l'espressione che non contraddice il Regolamento. Questo è ciò che spetta al Presidente. Esaminate gli interventi di oggi